una nota con la quale chiedevano di conoscere quali iniziative la Presidenza avesse intrapreso al fine di dare esecuzione agli esiti della votazione dell'Assemblea del pomeriggio di martedì. Chiedevamo altresì di conoscerne gli esiti nella consapevolezza e convinzione che, in ossequio alle nostre norme regolamentari, ma dico di più, all'articolo 64 della Costituzione, il Presidente del Consiglio fosse tenuto

non esiste più negli effetti del voto una differenziazione tra chi ha votato e chi non ha votato. L'Assemblea di Palazzo Madama aveva deliberato di invitare il Presidente del Consiglio a un dibattito sulla vicenda Telecom. Basta leggere gli atti parlamentari, la mia proposta, le modalità con cui ella ha messo in votazione quella nostra richiesta. Su questo credo non vi sia esigenza di approfondimenti né contraddizione alcuna. Un'ora dopo il voto - l'ho detto ieri - abbiamo letto con amarezza alcune dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Capogruppo della maggioranza che, con atteggiamento a dir poco inaccettabile, quasi a contestare il fatto che l'opposizione avesse fatto approvare quella richiesta di cambiamento del calendario, ribadivano che in funzione proprio di quel voto il Presidente del Consiglio sarebbe andato alla Camera e avrebbe disatteso - lo dichiaravano essi stessi - l'invito del Senato. una dichiarazione che abbiamo contestato ieri, che ancora oggi ci fa male e che preferiamo dimenticare, come preferiamo dimenticare le espressioni di chi ha pensato e ha accusato l'opposizione di voler trasformare quest'Aula del Senato in un pantano. Qui non c'è stato mai alcun pantano,

nel rispetto delle logiche di appartenenza e dei valori sui quali è fondata la nostra democrazia.

Ci saremmo attesi di più, signor Presidente, perché la sua appare una lettera - me lo consenta - ispirata ai doveri di ufficio, anche per la tempestività con cui ci è stata inoltrata; non possiamo che prenderne atto e apprezzarla sotto il profilo formale, ma non sotto il profilo sostanziale:

Non ci siamo. Con tutto il rispetto per il ministro Gentiloni, nei cui confronti non abbiamo nulla di personale, né di politico, il tema del dibattito era ed è diverso. Ci interessa sicuramente discutere della crisi finanziaria di una delle più importanti e strategiche aziende del nostro Paese, ma ci preme conoscere effettivamente come siano andati i fatti,

Da un lato abbiamo un Presidente del Consiglio che dichiara, *urbi et* *orbi*, di non sapere nulla di questa vicenda, dall'altro, collateralmente, vi è il suo consulente economico che mandava a Tronchetti Provera piani di dismissione e di nazionalizzazione dell'azienda. Chiediamo chiarezza su questi aspetti, sul pensiero del Presidente del Consiglio.

ci siamo vergognati di essere italiani, di essere rappresentati da quell'uomo in quel consesso, da quelle dichiarazioni!

perché il Presidente del Consiglio non va mai nei due rami del Parlamento a riferire. Vediamo, 9 ottobre 2001, sviluppi della situazione internazionale: presenza del presidente Berlusconi nei due rami del Parlamento; 7 novembre 2001, contingenti militari italiani all'estero: presenza del presidente del Consiglio Berlusconi nei due rami del Parlamento; 3 luglio 2002, omicidio Biagi: Berlusconi in entrambe le Camere; 25 settembre 2002, crisi irachena; 6 febbraio 2003, linee della politica estera italiana; 10 febbraio 2003, crisi irachena; 19 marzo 2003, crisi irachena; 12 novembre 2003, attentato a Nassiriya. Non ho finito: aprile 1997, questione albanese: presenza del Presidente del Consiglio dell'epoca, un certo professor Romano Prodi - credo sia lo stesso Presidente del Consiglio di oggi - in entrambi i rami del Parlamento; 26 marzo 1999, Kosovo: presenza del Presidente del Consiglio in entrambi i rami del Parlamento. dovrebbe ritrattare la sua dichiarazione di ieri: non solo non è convincente, ma è anche offensiva nei confronti della realtà storica della vita parlamentare.

un appello a lei che ci riserviamo (ove nel pomeriggio si dovesse realizzare questo strappo istituzionale) di rivolgere anche al Presidente della Repubblica. Vi è un precetto costituzionale da rispettare. Lo abbiamo citato più volte; la Costituzione vigente sta a cuore a tutti. È evidente che come lei è tenuto a rispettare e a fare rispettare il nostro Regolamento interno, il Capo dello Stato è tenuto, è garante - e di lui ci fidiamo - del rispetto dei precetti costituzionali. Non ci si venga a dire, da parte di taluni membri della maggioranza, che noi non possiamo imporre al Presidente del Consiglio una data e un'ora; non volevamo fare questo, non intendiamo farlo. Rientra nel *bon* *ton* istituzionale il principio delle intese, fa parte delle nostre regole; noi le conosciamo,

al Presidente del Consiglio l'individuazione del giorno, della data e dell'ora per realizzare il dibattito in quest'Aula. Abbiamo invece registrato toni piccati, a dir poco stizziti,

Signor Presidente, anch'io come il collega Schifani voglio partire dalla lettera che noi Presidenti dei Gruppi di opposizione le abbiamo mandato ieri sera. La sua risposta - per carità, cortese - ricevuta solo dopo pochi minuti mi ha fatto ritenere che anche lei abbia in qualche modo alzato le mani di fronte alla cocciutaggine del Presidente del Consiglio. Io spero, però, che in questi giorni lei abbia avuto modo, nel richiedere la presenza del Presidente del Consiglio a riferire in Aula, di ricordare allo stesso alcuni passaggi di questa inquietante vicenda. Com' è noto, l'11 settembre il Consiglio di amministrazione della Telecom si riunisce e comunica la decisione di scorporare da Telecom da Telecom la TIM creando due società. Martedì 12 e mercoledì 13 il presidente del Consiglio Prodi, che si trova in Cina, comunica di non sapere nulla sulla decisione assunta dal Consiglio di amministrazione Telecom nonostante

i giornalisti chiedono a Prodi cosa pensa della richiesta dell'opposizione di un chiarimento nell'Aula del Senato. Il

Domenica 17, Prodi è a Pechino dove dichiara che il Governo annuncerà martedì ai Capigruppo di Camera e Senato la propria disponibilità ad un'informativa urgente da parte di Ministri. Il 19 settembre, sempre il presidente Prodi, annuncia di essere disposto a riferire personalmente in Parlamento il 28 settembre, dieci giorni dopo, e avverte di essere disponibile ad andare in una sola Aula parlamentare.

Presidente del Consiglio, riferì l'8 aprile 1997 al Senato e il giorno dopo, il 9 aprile, alla Camera, quando informò deputati e senatori sulla crisi albanese.

sulla sicurezza del Papa, ma anche l'offesa continua che rivolge non solo ai senatori o ai deputati di opposizione ma all'Aula tutta. Signor Presidente, lei ha registrato il voto di quest'Aula e il Presidente del Consiglio non può disattendere quel voto. Non è assolutamente pensabile Non è assolutamente pensabile che questo accada. Pertanto, alla luce di quanto accaduto ieri - gli arresti di Milano legati in qualche modo alla vicenda Telecom -, poiché credo

partiti politici, ma credo debba farlo anche lei, presidente Marini, perché l'imbarazzo è di tutti ma quello più grande, per quanto riguarda questa vicenda, deve essere proprio il suo per come viene trattata questa Aula del Parlamento da parte del Presidente del Consiglio. Dopo l'intervento sui lavori del Senato del senatore Schifani, si è aperta una discussione politica su un fatto rilevante.

chiedendo all'Assemblea di proseguire i lavori per la quale stamattina essa è stata convocata, cioè la discussione generale sull'ordinamento giudiziario.

di civiltà assoluta. Quindi apprezzo che due autorevoli Capigruppo dell'opposizione facciano in Aula questo richiamo.

necessità che venga personalmente il Presidente a riferire. Credo che oggi pomeriggio si svolgerà un dibattito esauriente su tutti gli aspetti che lei ha richiamato e che il Ministro delle comunicazioni, per incarico del Governo, potrà

Presidente Matteoli, il presidente Berlusconi - cito il presidente Berlusconi perché era il capo della maggioranza nella passata legislatura ed è il capo della coalizione della quale anche lei e la sua formazione politica fate parte - nella passata legislatura non ha mai partecipato alle sedute della Camera dei deputati sul *question time*. Chiamato ripetutamente non ha mai una volta, nonostante un'esplicita previsione del Regolamento, partecipato. *(Ulivo)*. Più volte il presidente Berlusconi - e tutti i parlamentari lo ricordano - ha dichiarato di considerare i lavori d'Aula del Parlamento una perdita di tempo. espressioni testuali usate dal presidente Berlusconi. Penso che dobbiamo considerare tutte queste circostanze. Amici senatori, penso che dobbiamo tenerle ben presenti. Nel momento in cui vogliamo - come tutti vogliamo - mantenere il dibattito su una cifra di civiltà e di rispetto reciproco, dobbiamo cercare di svolgere il nostro lavoro seguendo quanto più possibile

Grazie

poco più di una giornata alla settimana. Noi stiamo usando questo poco tempo disponibile per discutere d'altro. Oggi abbiamo un intero pomeriggio per discutere la questione

Presidente, per rispetto nei confronti dei colleghi cerco sempre di ascoltarli attentamente. Ho ascoltato attentamente anche il collega Zanda e vorrei partire proprio dalle sue considerazioni.

della vicenda in sé ed entrano in gioco i rapporti istituzionali tra poteri e tra istituzioni dello Stato. Questo è il dato fondamentale sul quale vorrei porre l'attenzione; altrimenti sarei costretto a ripetere le parole del presidente Schifani e del presidente Matteoli, che condivido pienamente e faccio mie. Vorrei quindi porre l'attenzione su un'altra questione, signor Presidente, e mi rivolgo direttamente a lei. io credo che questi mesi di frequentazione siano stati improntati al massimo rispetto e, se mi consente, anche a tratti di cordialità. È quindi con il massimo rispetto verso di lei e, sempre se mi consente, con qualche tratto di cordialità che vorrei porre l'attenzione su alcuni punti della lettera che lei, così tempestivamente e cortesemente ha voluto inviarci in risposta alla nostra sollecitazione. Vorrei citare testualmente. Lei ci dice: «Le comunico che fin dalla serata di ieri, immediatamente dopo il voto del Senato, ho provveduto ad informare i Ministri competenti e la Presidenza del Consiglio della decisione assunta dalla maggioranza dell'Assemblea. A conclusione dei miei contatti le comunico che verrà il ministro Gentiloni». Mi scusi, signor Presidente, ma lei non ha seguito altro che

caso c'è stato un voto dell'Aula, c'è stato un caso politico che ha occupato l'attenzione di tutti i *media* e che ha interessato l'opinione pubblica. C'è stato un Senato che

le chiedo di fare, anche in queste ore, tutto il possibile e di mettere in atto le azioni straordinarie che questa votazione, che ha carattere straordinario, si merita. Questo è il dato fondamentale. Altrimenti è evidente che lei non ci protegge, non protegge la dignità del Senato nella misura in cui ci aspettiamo debba essere protetta. Vorrei veramente che lei meditasse su tale questione.

non so cosa potrà dirci. Ci parlerà del piano frequenze? Ci parlerà della telefonia fissa? Di cosa ci parlerà? Non so, non ha nessuna competenza sui problemi odierni, che sono: che fine farà la Telecom sul piano finanziario e industriale e come mai, guarda caso, non appena è cambiato l'amministratore delegato, scattano degli arresti a Milano proprio su tale questione. Sarà un caso, può darsi, capirete che è un caso abbastanza curioso, anche perché «Il Sole 24 Ore» ieri preannunciava di fatto questi arresti. Basta leggere tra le righe l'articolo che «Il Sole 24 Ore» scrive a proposito dell'attività dei pubblici sarebbe successo qualcosa molto a breve. Sono tutte questioni sulle quali credo che il ministro Gentiloni non abbia proprio nulla da dirci. Quindi lascio liberi i senatori di venire o meno; io non verrò sicuramente, non certo per mancanza di rispetto, ma perché - come diceva giustamente il collega Zanda - abbiamo molte cose da fare, il tempo è tiranno e io cercherò di utilizzarlo meglio. Un suggerimento potrei avanzarlo, signor Presidente, per quanto riguarda il presidente Prodi. Lei l'altro giorno ci ha detto che non poteva mandare i carabinieri a prenderlo; è vero: provi a mandargli le guardie svizzere.

sulla richiesta da parte del Senato al Governo di essere presente in Aula con la conseguenza che il Governo è libero di scegliere da chi farsi rappresentare. la vicenda fosse stata impostata in questi termini, così come lo era stata circa un mese fa, non avrei avuto alcun dubbio nel dire che il Governo decide da chi farsi rappresentare.

UDC - della sua assoluta volontà di dar seguito alle deliberazioni del Senato, vorrei evitare che si commetta l'errore di ritenere che noi abbiamo chiesto la presenza del Governo. Se noi avessimo chiesto questo, il Presidente del Senato chiederebbe al Governo da chi intende essere rappresentato. Ma possiamo noi chiedere questo? proposito, ho il timore che l'articolo 59 del Regolamento, che ci legittima a far questo e che è attuativo di una norma costituzionale, che espressamente, e giustamente, ritiene che questo si possa fare, non sia stato sufficientemente considerato. L'articolo 59 del nostro Regolamento, così come l'articolo 64 della Costituzione, stabiliscono che il Senato chiedere la presenza non del Governo, ma di «rappresentanti del Governo» o di «membri del Governo». Ciò perché il sindacato ispettivo, che è un punto fondamentale del regime parlamentare, si esercita con l'atto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e con la richiesta di presenza, individualmente considerata. È ovvio che all'interrogazione può rispondere un altro esponente del Governo perché l'interrogante può aver sbagliato nell'identificazione del responsabile; è ovvio che all'interpellanza può rispondere un altro soggetto, perché l'interpellante può aver sbagliato nell'imputazione della responsabilità. Tuttavia, quando si chiede la presenza del Presidente del Consiglio questo errore non è più possibile, perché qualunque Ministro può non essere specificamente responsabile degli atti del Governo, ma non il Presidente del Consiglio, che per Costituzione è responsabile complessivamente non degli atti giuridici, ma degli atti politici compiuti da tutti i Ministri. Invito ancora una volta il

ma abbiamo il diritto di chiedere che «quella» persona venga, non che venga il Governo nella sua generica composizione. Ritengo che il Presidente del Senato sia specificamente autorizzato dal nostro voto a far capire e a dire al Presidente del Consiglio che o viene lui, e sceglie la data in cui venire e non è tenuto persino a parlare, o non può mandare un altro che non può essere legittimato a rappresentare se non sé stesso e il Governo; non c'è in tal caso la rappresentanza del Presidente del Consiglio specificamente richiesta dal Senato. È una questione di estrema delicatezza.

essere esponente del Governo mandato dal Governo stesso in Parlamento e si poteva innestare una polemica politica sulla sufficienza della sua presenza, ma oggi c'è un problema di legittimità,

il 28 settembre alla Camera, fare presenza, avrebbe risolto il problema anziché affrontare una questione del genere. Penso che lui che ha un consigliere economico così avveduto come Rovati, forse non ha un consigliere giuridico sufficientemente scaltro. Non lo so, questo è un problema di organizzazione della Presidenza del Consiglio. Dal punto di vista istituzionale il Presidente del Senato non è latore di una richiesta dell'Aula del Senato al Governo perché sia presente. Il Presidente del Senato è latore di una richiesta al Presidente del Consiglio, domani potrebbe esserlo al Ministro dell'agricoltura, dei trasporti o degli esteri, perché il Senato ha il diritto, in base alla Costituzione, di chiedere che una persona specifica venga e la persona può decidere quando venire. Mi permetto di insistere su tale questione, signor Presidente.

coprire la responsabilità del singolo Ministro ponendo la questione di fiducia dell'intero Governo. Quindi, ritenevo la questione ammissibile allora ed è ammissibile oggi. Ma, ancora una volta, ritengo che oggi il Presidente del Senato debba ribadire al Presidente del Consiglio che non può mandarci un'altra persona. deve soltanto dire al Presidente del Senato: «Visto che ho l'obbligo di assistere e non di parlare, adempio all'obbligo nel giorno... e il e il Presidente del Senato ci dirà: «Il Presidente del Consiglio verrà il giorno...» e la nostra richiesta, costituzionalmente vincolante per il Presidente del Senato come per il Presidente del Consiglio, diverrà

Nella mia brevità voglio però sottolineare alcune questioni delle quali abbiamo parlato ieri nell'incontro dei Capigruppo della minoranza. Con la sensibilità di un cittadino italiano

con semplice sensibilità politica ma che sono iscritte nel nostro Regolamento e nella nostra Costituzione. Mi riferisco alla possibilità, alla necessità e all'obbligo per chi chiamiamo

il senatore Cutrufo, il senatore D'Onofrio, il senatore Schifani o il presidente Marini, che comunque è il presidente del Senato della Repubblica. noi siamo stati eletti, sempre che siamo ancora nel sistema che conosciamo, quindi un sistema democratico, parlamentare e bicamerale. In tale sistema si dice appunto

peraltro, rispetto a quella del Senato, di tipo generico, come può essere impropriamente definita - e la risposta negativa ad una chiamata del popolo italiano. Noi infatti siamo il popolo italiano nel momento in cui interloquiamo da questi microfoni in quanto eletti

al Senato), chiede al Presidente del Consiglio di conferire su un argomento di tanta importanza e rilevanza, che occupa da più di una settimana le prime pagine di tutti i giornali italiani e internazionali. ripeto, con un voto; quindi, c'è un voto del popolo italiano a maggioranza in Senato che chiede tale presenza e c'è un rifiuto del Presidente del Consiglio, eletto dallo stesso popolo poco tempo fa, a venire a riferire.

ma in questo caso, di fronte ad un rifiuto al popolo italiano di venire a conferire nella Camera alta del Parlamento, cosa è previsto dalla Costituzione?

strumentalizzare dal punto di vista politico; c'è invece un'esigenza legittima del popolo italiano di sapere dal Presidente del Consiglio cosa sta accadendo nella vicenda Telecom.

da quella parte economica che aspetta provvedimenti come il cuneo fiscale e tanti altri. C'è un grido di dolore nel popolo italiano, che vede disattese anche le sue richieste di colloquio

Presidente, ritengo assolutamente legittima l'iniziativa assunta dall'opposizione anche questa mattina, non solo per i toni usati, ma anche e soprattutto ma anche e soprattutto per gli argomenti che sono stati portati alla nostra attenzione, anche se secondo me alcune

all'accusa che le è stata rivolta di non avere ottemperato a quanto previsto dalla Costituzione essendo stata richiesta espressamente la presenza in Aula del Presidente del Consiglio. Ritengo, Presidente, che lei abbia agito con grande linearità, facendo tra l'altro quello che aveva già preannunciato in Aula, cioè chiedere al Governo di essere presente a seguito di una decisione dell'Aula. Certamente, l'opposizione fa il suo mestiere, dal punto di vista politico ed istituzionale e nel confronto parlamentare.

contenuto, c'è una differenza, che dev'essere tenuta in considerazione, tra una legittima richiesta politica, magari a seguito di affermazioni rese dal Presidente del Consiglio che non si condividono,

sul piano politico, sia per le responsabilità politiche che l'opposizione ritiene di avere nei confronti del Presidente del Consiglio, sia per quanto riguarda lo sviluppo

chiudere questa prima fase del confronto, che si svilupperà ulteriormente con la presenza del primo ministro, l'onorevole Prodi. *(Applausi

l'assetto industriale del Paese su un punto così delicato, qual è quello delle telecomunicazioni. Una minoranza sceglie le modalità con cui

si auspicava la presenza del Presidente del Consiglio. Credo che il Presidente del Senato non abbia potuto fare altro che chiederla e riceverne la risposta che qui

sugli assetti proprietari di Telecom, che non sono non significativi in un Paese che dovrebbe ripensare - e anche negli atti del Governo lo fa - un'idea di politica industriale; e non può esserci, come tutti sappiamo, una politica industriale se non c'è una politica nel settore telecomunicazioni. Per questo, credo

svolgere solo poche considerazioni. Ho chiesto d'intervenire perché credo che i toni con i quali stiamo discutendo questa mattina dovrebbero essere quelli con i quali abitualmente il Senato della Repubblica dovrebbe discutere di tutto.

perché nei mesi e negli anni precedenti, probabilmente, vi era stata una messa in discussione, anche se non suffragata da alcuna modifica costituzionale, della centralità del Parlamento, del parlamentarismo del nostro sistema costituzionale. Sono ben lieto quindi che su una questione delicata vi sia stato, da parte degli amici delle opposizioni, il recupero di una valenza parlamentare piena che ha consentito al Senato di indicare con fermezza attraverso un voto quali potessero essere i momenti di un percorso di chiarimento su una vicenda che ha interessato l'opinione pubblica complessiva. ben lieto che vi sia stata un'inversione di tendenza anche culturale rispetto alla pratica costituzionale della Casa delle Libertà che, ripeto, in passato, attraverso i suoi massimi esponenti, aveva anche considerato le venute in Parlamento

(lo ricordo a me stesso) è che, rispetto ad un presunto o lasciato intendere rifiuto di sottoporsi ad un dibattito parlamentare, i fatti sono maturati in modo tale che, al di là delle appartenenze di maggioranza o minoranza, vi sono state prese di posizione che hanno determinato il convincimento che fosse giusto che la questione venisse affrontata in modo corretto nel Parlamento della Repubblica. Si tratta di un passo avanti; anche i comportamenti e le prese di posizione dei partiti dell'attuale maggioranza hanno fatto sì che ciò sia potuto avvenire. Ritengo che se continuiamo su questa strada tutto il Parlamento ne guadagnerà. Ringrazio il presidente Marini perché ci ha consentito di arrivare a ciò,

è *bon ton* istituzionale consentire ai senatori di partecipare ai vari livelli di discussione politica. Con questo non vogliamo minimamente incidere sui lavori d'Aula. Ovviamente, saremo un po' compressi compressi nelle nostre facoltà, se ci dovessero essere momenti di decisionalità ai quali noi, senatori dell'Italia dei Valori, non dovessimo poter partecipare a causa di calendarizzazioni di molto antecedenti a ciò che è avvenuto l'altro ieri. Quindi, molto dimessamente, sottopongo all'Aula e al presidente Marini anche tale esigenza dei senatori dell'Italia dei Valori. Vorrei concludere il mio breve intervento rimarcando ancora una volta

della discutibilità della fissazione di una data precisa (perché queste cose si risolvono con il consenso nel rapporto con il Governo in generale o con il Presidente del Consiglio), mi sono

che è un fatto a sé), il Presidente del Consiglio ha indicato, assumendosene le responsabilità politiche, un Ministro a rappresentarlo. Oggi qualcuno ha ricordato nel dibattito

Su questo punto, che è una novità rispetto all'ordine del giorno approvato, mi riservo di svolgere l'azione che il Presidente del Senato deve svolgere,

all'Aula qual è la situazione che si è determinata. Poi si torna alla politica; non so e non credo che vi siano strumenti al di là della convinzione per imporre una decisione

anche se non fanno parte del Senato, hanno il diritto e anzi l'obbligo di partecipare alle sedute, se richiesti, dell'Aula. PRESIDENTE. Senatore Divina, abbiamo discusso per un'ora di questo punto quindi non credo che al Regolamento o alla Costituzione si possa aggiungere alcunché.

L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*bis*, n. 1, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano,

Il 28 febbraio 2005, il collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della nostra Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*. Il tutto in relazione a vicende concernenti la nomina degli amministratori giudiziali nella procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ELDO SpA e della società ELDO SpA dell'ottobre del 2002. Nei confronti di Antonio Marzano, il collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, dopo una prima attività istruttoria, dispose, in data 27 settembre 2004, l'archiviazione in relazione al reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale - parliamo di ipotesi

di reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale. La procura della Repubblica di Roma, in conseguenza delle risultanze di ulteriori attività di indagini svolte, in data 22 novembre 2004, ha trasmesso al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma richiesta di procedere per il reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale nei confronti del ministro per le attività produttive *pro tempore* Antonio Marzano. Con nota del 23 gennaio 2006, la procura della Repubblica di Roma ha richiesto al collegio per i reati ministeriali che, esclusi i presupposti per disporre l'archiviazione, si trasmettessero gli atti al suo ufficio per la loro successiva rimessione al Presidente del Senato affinché venisse concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro *pro tempore* Antonio Marzano, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Nella relazione il collegio per i reati ministeriali, dopo essersi diffusamente soffermato ed aver concluso in senso positivo circa il tema della utilizzabilità dei verbali delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) sulla base delle quali l'ufficio del pubblico ministero aveva proceduto alle contestazioni, ha ritenuto condivisibile, anche alla luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie effettuate dal collegio medesimo, la richiesta dell'ufficio del pubblico ministero di avanzare alla Camera competente richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'allora ministro *pro Alla luce di tutte le risultanze istruttorie, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che, pur mancando la prova diretta di un intervento dei privati sulla persona del ministro Marzano

il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che, pur mancando la prova diretta di un intervento dei privati sulla persona del ministro Marzano (significa che, pur non essendoci alcuna prova che nessuna delle persone poi nominato commissario liquidatore abbia parlato con il Ministro) devoluta alla discrezionalità del Ministro - resta la convinzione che la scelta operata da quella nomina e quindi dei commissari non sia stata assolutamente improntata a criteri di stretta discrezionalità, ma sia stata orientata in favore dei soggetti segnalati anche dallo stesso imprenditore. Il Collegio per i reati ministeriali ha quindi analiticamente esposto le ragioni per cui ritiene che ricorrano in concreto, nel caso in esame, gli elementi necessari ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 323 del codice penale, muovendo dall'assunto che ben può ben esservi spazio per la configurabilità del reato ipotizzato, ove la norma che impone al pubblico ufficiale scelte imparziali sia stata concretamente violata con la scelta di un soggetto che non viene individuato per le sue caratteristiche, professionali. In conclusione, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che, qualora le nomine in questione siano state finalizzate solo ad interessi privati, sia prefigurabile l'ipotesi di violazione dell'articolo 323 del codice penale. Questa è la costruzione che, attraverso la richiesta sostenuta dal tribunale per i Ministri, viene sottoposta alla Giunta. La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 5, 6, 11, 12, 18 e 19 luglio 2006, dando conto, proprio per la delicatezza della vicenda, di un approfondimento che era un atto dovuto. Nel corso dell'audizione, il professor Marzano ha riepilogato i termini della vicenda, che ebbe inizio nel novembre 2001 su iniziativa della procura della Repubblica di Potenza: questa formulò a suo carico, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive, un'ipotesi di corruzione in relazione alla nomina degli avvocati Giovanni Bruno e Roberto Marraffa come commissari straordinari di società in amministrazione straordinaria. Dopo una declaratoria di incompetenza del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Potenza - abbiamo visto anche attualmente procure che si dichiarano competenti a tutto tondo sul territorio nazionale e poi questa competenza viene viene meno - il procedimento venne trasferito a Roma. Il 27 settembre 2004 il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma dispose l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti, sottolineando innanzitutto che la maggior parte del materiale probatorio su cui si fonda la nuova ipotesi accusatoria è costituito da intercettazioni ammissibili ma che comunque le persone sottoposte ad intercettazioni telefoniche venivano definite nel precedente provvedimento di archiviazione come avvezze alla menzogna e alle allusioni. Un altro profilo sul quale secondo il professor Marzano deve essere richiamata l'attenzione è quello attinente alla natura dei poteri attribuiti al Ministro dal decreto legislativo n. 270 del 1999, con specifico riferimento alla nomina dei commissari giudiziari e dei commissari straordinari nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal medesimo decreto. In particolare, la designazione dei commissari giudiziali è operata dal Ministro su richiesta del tribunale che deve procedere alla dichiarazione dello stato di insolvenza ed è un atto rimesso alla discrezionalità del Ministro.

che seguiva ad una dichiarazione di uno stato di insolvenza da parte del tribunale. Quindi, a monte, l'*input* non partiva da lui e comunque la regolamentazione esistente prevede una discrezionalità totale in capo al Ministro nella individuazione dei professionisti che devono essere nominati. A diversi quesiti, il professor Marzano ha replicato dichiarando che l'assenza di previsioni regolamentari - la Giunta, infatti, ha chiesto come mai

ha anche ribadito che a più riprese, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Ministro delle attività produttive, sollecitò il Ministero della giustizia allo scopo di pervenire finalmente all'adozione dei regolamenti in questione, obiettivo che però, per svariate motivazioni, non fu possibile raggiungere Prescindendo da qualunque valutazione di merito della richiesta di autorizzazione a procedere in ordine alla sussistenza o meno delle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la Giunta ritiene opportuno richiamare l'attenzione su un profilo di ordine processuale che appare dirimente. Esso è rappresentato dall'individuazione dei presupposti che, ad avviso del Collegio per i reati ministeriali, legittimerebbero una decisione di archiviazione. Il Collegio ritiene che «la richiesta di autorizzazione si pone esclusivamente come alternativa procedurale alla decisione di archiviazione alla quale il tribunale può ricorrere esclusivamente a fronte di notizie palesemente prive di fondamento, e non implica perciò una valutazione nel merito delle accuse». Secondo la Corte costituzionale, invece, il Collegio inquirente è dotato di un potere di indagine eccezionalmente ampio, il cui esercizio è funzionale ad una doppia valutazione di merito: quella spettante allo stesso Collegio inquirente (che può disporre l'archiviazione), e quella, invece, di richiedere l'autorizzazione a procedere, quindi collegata a un potere delle Camere di negare o concedere l'autorizzazione a procedere. quel Collegio non esercita appieno i limiti precisi del suo potere e non archivia una situazione rispetto alla quale indica degli elementi che dovrebbero portare all'archiviazione, rimette alla Giunta una valutazione che sarebbe oltre quelli che la Costituzione prevede come i confini fisiologici. È agevole, quindi, concludere come una corretta interpretazione logico-sistematica sostenga il disposto del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, che attribuisce alla "archiviazione" prevista dalla legge costituzionale contenuti più ampi di quelli previsti dal codice di rito vigente. La normativa recata dalla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 affida pertanto al tribunale per i Ministri il potere-dovere di delineare in modo preciso e puntuale la fattispecie di reato contestata in concreto agli imputati, sulla base di riscontri indagativi ampi e completi, all'acquisizione dei quali sono funzionali i poteri istruttori eccezionalmente ampi di cui il tribunale medesimo è investito: solo l'assolvimento di tale compito consente al Senato di procedere ad una verifica effettiva circa l'eventuale sussistenza delle finalità previste dal terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale citata. Al contrario, nel caso di specie, la prospettazione compiuta dal Collegio per i reati ministeriali come evidenziato singolarmente restrittiva in ordine ai presupposti dell'archiviazione - costringerebbe la Giunta - e quindi, di conseguenza, l'Aula - a operare le proprie valutazioni sulla base di risultanze istruttorie per definizione incomplete. La modestia della cognizione di competenza della Giunta impedisce di riversare sul Parlamento le conseguenze di un comportamento omissivo da parte del Collegio, il quale, tra l'altro, espressamente dichiara che manca la prova diretta del collegamento tra i coindagati e il ministro *pro tempore* Antonio Marzano. Occorrerà quindi che il Collegio valuti se si è davvero in presenza di un'ipotesi accusatoria dotata di un ragionevole margine di fondamento, sulla base di riscontri indagativi ampi e completi che consentano al Parlamento di esercitare il proprio potere valutativo.

affinché il Collegio non si limiti ad escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato, ma decida o per l'archiviazione o per la presenza di un'ipotesi accusatoria autonoma e dotata di fondamento. *(Applausi

documento della Giunta, volto che la Giunta ha concluso i propri lavori e il proprio incarico - come or ora ha ricordato il relatore, senatore Manzione - con una decisione unanime, che peraltro, lo dico da garantista, quale mi sento e sono, non è sfavorevole nei confronti della persona interessata dai fatti che sono contestati, cioè il professor Marzano. Marzano. Rimedierò a questa inusualità del mio intervento con la brevità dello stesso. Spiego subito perché mi sono risolto, tuttavia, ad intervenire. Lo faccio premettendo che non posso e non si può non riconoscere e credo che ne debba rimanere traccia oggettiva nei lavori di questa mattinata - l'eccezionale qualità del lavoro svolto della Giunta, sia con riferimento al documento proposto dal relatore, senatore Manzione, sia con riferimento alla relazione che egli ha svolto in Aula, in qualche misura di sintesi e quindi di riduzione della grande articolazione che viceversa connota il documento, e, d'altra parte, di esplicazione

Per quanto riguarda la normalità, credo che la stessa risieda in quanto anche il relatore Manzione ha incidentalmente ricordato e in quanto si apprende dalla lettura del documento che ci è proposto. con un'inchiesta da parte del procuratore della Repubblica di Potenza, a cui fa subito seguito una dichiarazione di incompetenza di quel procuratore a conoscere la vicenda. È argomento che ci sta inseguendo nelle cronache giornalistiche ormai da anni, senza che nessuno, dentro e fuori quest'Aula, dentro e fuori il Palazzo dei Marescialli, dove ha sede il Consiglio superiore della magistratura, prenda una posizione ferma sul punto. Al contrario, fra poche decine di minuti noi affronteremo un disegno di legge che, fra le altre sue finalità, ha quella di sospendere un decreto legislativo che ha introdotto nel nostro ordinamento ordinamento la possibilità di un processo disciplinare nei confronti del magistrato, caratterizzato da precetti di tipizzazione, di tipizzazione, dalla obbligatorietà dell'azione e dalla possibilità di introdurre sanzioni effettive non contro il magistrato, ma nei confronti di quel magistrato che manca ai suoi doveri verso la collettività. Vede, signor Presidente, l'avere una procura della Repubblica avviato e condotto un'inchiesta essendo palesemente incompetente a farlo, come non il senatore Caruso, non l'uomo politico, non altri, non il giornale, ma altri giudici hanno seccamente ed inequivocabilmente stabilito anche in questa occasione, al di là di quanto determina nei confronti personali del destinatario dell'inchiesta - al professor Marzano non ha certo giovato e fatto piacere la conduzione della stessa determina conseguenze su cui non ci si può non interrogare in ordine alla possibile rilevanza disciplinare. Avviare un'inchiesta penale, da parte di una procura, vuol dire occupare risorse umane, del giudice stesso e dell'apparato che è intorno al giudice; questo vuol dire recare discapito ad altre indagini e ad altro contrasto criminale, che rientrano nei doveri di quel giudice e nelle aspettative dei cittadini nei confronti di quel giudice. Vuol dire occupare le risorse della polizia giudiziaria, che il pubblico ministero controlla non come una sua dotazione personale, ma per l'esercizio di un dovere di oculato uso di una risorsa dello Stato che ha particolare carattere di delicatezza. Vuol dire occupare risorse economiche quando su quotidiani e nel corso di interviste televisive si ascoltano i procuratori generali della Repubblica e i presidenti di corte d'appello lamentare, forse in maniera esagerata ma altre certamente con fondamento, la mancanza dei mezzi e delle risorse materiali più elementari. Vuol dire determinare quell'allungamento dei tempi del processo in generale, quella lentezza della giustizia che nessuno manca di declamare come iattura che ha colpito il nostro Paese e da cui esso non riesce a liberarsi, ma poi nulla fa perché tutto ciò sia impedito. Direi che la vicenda del professor Marzano su questo

Tanto la liquidazione coatta amministrativa quanto le amministrazioni straordinarie si caratterizzano nel panorama delle procedure concorsuali come procedimenti non a carattere esclusivamente giudiziario, ma a carattere prevalentemente amministrativo. La prevalenza amministrativa si connota anche nel fatto che chi è alla guida di queste procedure mirate al risanamento delle aziende in crisi non è un soggetto nominato dal giudice con fini liquidatori, ma un soggetto nominato dal Ministro. Signor Presidente, la gestione delle liquidazioni coatte amministrative e delle amministrazioni straordinarie nel nostro Paese ha costituito uno scandalo vero fino a quando non ha assunto l'incarico di ministro il professor Marzano.

posizioni parassitarie che erano state formate per non guidare queste aziende e queste situazioni procedurali fallimentari a tutto danno dei creditori.

che a distanza di decenni non hanno visto chiusi gli stati passivi di liquidazione coatta amministrativa e le amministrazioni straordinarie da parte di commissari giudiziari e di commissari liquidatori virtuali virtuali nominati in precedenza e avvicendati dal ministro Marzano. Con buona pace di tale dottor Visconti, che leggo essere stato il predecessore del funzionario addetto alle nomine dei commissari giudiziari, che si lamenta del fatto che il ministro Marzano abbia modificato i sistemi di nomina, forse assumendosi qualche responsabilità in più, che oggi è chiamato a pagare, è stato eliminato in tutta evidenza il sistema della proposta, che aveva portato sistematicamente i soliti noti al vertice delle procedure concorsuali di quel tipo per incassare pingui compensi e per non fare mai assolutamente nulla. prudenza del ministro Marzano, sempre nelle pieghe di questo documento si dice che egli riceve attraverso terzi, perché il tribunale stesso riconosce che non ha mai avuto rapporti con questi tali, varie proposte di nomina. Alla fine - conclude il tribunale - due dei soggetti nominati corrispondono a quelli che erano sollecitati dall'imprenditore del caso. Due su tre,

una modifica volta al raggruppamento dei due ordini - dunque una figura istituzionalmente e ontologicamente indipendente. Siccome quello dei commissari giudiziari è un collegio perfetto che che funziona solo se sono in tre e solo se si esprime una maggioranza, va da sé che la condotta del ministro Marzano in questa vicenda mi sembra non solo improntata alla sua generale volontà - che egli ha orgogliosamente richiamato nella sua audizione alla Giunta - di modificare uno stato di cose indecente, ma anche a grande prudenza. Presidente, ha ricordato quello che è il passo significativo dell'ordinanza del tribunale per i Ministri. Tale tribunale dice che non vi è una prova al mondo che vi sia stato un contatto diretto tra il ministro Marzano e le persone che egli ha nominato

pianeta Marte. È assolutamente fisiologico ed evidente che chi vuole essere nominato, chi aspira a queste nomine per proprio interesse, ambizione o per qualsiasi ragione al mondo, solleciti questa sua nomina e che quindi al Ministro pervengano delle richieste, come è avvenuto nel caso dei due commissari giudiziari poi nominati. Il

è documentalmente professionista di grande vaglia e su cui la capacità di espressione discrezionale della propria decisione del ministro Marzano certamente non ha fallito nel merito. La Giunta

e mi avventuro consapevole in un terreno che non è mai stato specificamente il mio - il dovere della nostra Giunta sia in questa occasione quello di fare un passo in più

Manzione di riflettere su questo punto, anche nella sua intrinseca coerenza. Il tribunale per i Ministri non può con la mano destra dire che non c'è una prova al mondo della fondatezza della notizia di reato e con la mano sinistra chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Marzano. Ma procedere a che cosa? Per l'accertamento di che cosa? Per pervenire a quale risultato? Credo, signor Presidente, che il Senato farebbe buon servizio, non al professor Marzano, ma alla necessità di chiudere vicende che sono partite con il piede sbagliato del procuratore della Repubblica di Potenza e che rischiano di arrivare con il piede altrettanto sbagliato in un processo inutile, in un pletorico e inutile utilizzo delle risorse dello Stato. Chiedo al relatore - non è una proposta che avanzo all'Aula, ma al relatore - di modificare la sua proposta chiedendo che questo affare ritorni presso la Giunta perché essa possa riesaminarlo in un'ottica più coraggiosa,

grave reato che sarebbe stato commesso dagli uffici del ministro Marzano, e da lui in particolare, è il seguente. Il primo documento ritrovato è il *curriculum vitae* dell'avvocato Bruno, che appare redatto su carta intestata del predetto. Esso reca l'intestazione di ricezione del *fax* in data tal dei tali e sembra poi trasmesso, quale documento, al Ministro, affinché questo possa operare le scelte che, in perfetta discrezionalità, la legge gli consente di effettuare. Ora, mi meraviglio profondamente quasi provo un senso di ridicolo nel pensare che un *curriculum vitae* non debba essere redatto e sottoscritto dalla persona interessata, che presenta se stesso, le proprie caratteristiche, i dati anagrafici sua professionalità per far capire a colui che deve decidere di essere in grado di espletare un determinato incarico. Eppure i tribunali, i giudici e i magistrati lo considerano tra le prove essenziali di questo abuso, di questo sopruso, di questo atto disonesto. Sono profondamente e sempre più meravigliato, e a volte mi meraviglio di meravigliarmi, che noi a volte si debba continuare a perdere il tempo del popolo italiano che ci manda qui a rappresentarlo per sviscerare questioni soltanto burocratiche che partono da cause politiche di politicanti, non di uomini politici, che cercano di utilizzare con ogni mezzo il loro potere, o il presunto loro potere, per minare i meccanismi di un Governo che cerca e ha cercato, facendo anche con buoni risultati il bene del Paese, di migliorare la condizione dei cittadini. Forse spesso dimentichiamo che siamo qui tutti, come ha ricordato il senatore Cutrufo, perché rappresentiamo il popolo italiano. Ricordo che da bambini, durante le feste di paese, ci si divertiva a mettersi di fronte alla banda che suonava gli ottoni masticando metà limone per far in modo che le smorfie provocate

commissari. Ricordiamoci, per esempio, l'eterno e mai risolto problema, che ormai si è incancrenito, dei commissari che dovrebbero ripulire la Campania dai rifiuti: nessuno è mai andato a verificare cosa stiano facendo, come abbiano utilizzato i fondi e perché i Comuni non abbiano pagato le ditte che hanno vinto le gare di appalto. Ciononostante, in quest'Aula, per tante volte, siamo stati a chiamati a rifinanziare con decine di milioni di euro l'assoluta mancanza di professionalità. I casi allora sono due: o questi signori sono degli incapaci o sono chiaramente dei ladri. Lo abbiamo già detto, ma non succede niente. Stiamo ora andando a fare le pulci ad un Ministro che ha avuto l'ardore di utilizzare, tra le altre cose, il *curriculum vitae* di un avvocato, il quale, parlando di se stesso, attesta di essere in grado di espletare il suo incarico.

Sia ieri che oggi, abbiamo cercato di capire come mai un Presidente del Consiglio eletto dagli italiani non vuole parlare con gli italiani, non vuole venire in Senato a parlare con noi che siamo l'espressione del popolo. In particolare, i miei colleghi ed io siamo l'espressione del popolo del Nord che non lo ha votato e saremmo anche curiosi di sapere

Si parla anche di intercettazioni e non si sa se ci sia un legame, ma sicuramente ci sarà qualcosa di più importante del *curriculum vitae* di un avvocato che vuole fare il commissario

*(FI)*. Presidente, credo sia doveroso intervenire su questo tema, ancorché la Giunta le elezioni e immunità parlamentari abbia deliberato all'unanimità su quanto illustrato dal relatore, collega Manzione, sulla base di una relazione scritta molto articolata

per eventuali successive iniziative analoghe che potessero verificarsi nel futuro.

ma è una conclusione responsabile, che tiene conto del contesto normativo nel quale si pone questa vicenda

concessione o dal diniego dell'autorizzazione a procedere allo stato degli atti, così come consegnatici dal tribunale dei Ministri. Qual è il punto?

ma manca l'oggetto del delitto. È come se incriminassimo qualcuno per omicidio, ma la vittima non fosse stata nemmeno individuata, scoperta e riscontrata. Così è avvenuto in questa vicenda: vi è un procedimento a carico di un Ministro e, al di fuori di qualsiasi dimostrato o dimostrabile collegamento con certi personaggi, qualcuno ha millantato un certo credito; manca, però, qualsiasi elemento, anche indiziario, che colleghi il Ministro a questi personaggi. signor Presidente e colleghi, la legge che disciplina i procedimenti

non impedisce all'autorità giudiziaria inquirente, una volta ricevuta la *notitia criminis*,

almeno un *fumus* di sussistenza. Anzi, è necessario che vi sia un minimo di indagine preliminare e, probabilmente, anche l'espletamento della stessa,

venire denegata o meno) sulla base del fondamento di un interesse pubblico al verificarsi di quel comportamento ipotizzabile come reato. reato. Se non vi è, dunque, un minimo di analisi, di approfondimento, di istruttoria sugli elementi del reato, della fattispecie criminale, com'è possibile, alla Giunta e all'Aula, valutare se sussista l'interesse pubblico, laddove non è nemmeno provato, o comunque fondato, il fatto criminoso addebitato o addebitabile al Ministro in tale particolare situazione? Per questo la Giunta chiede all'Aula di rinviare gli atti

ma perché probabilmente non ha avuto la volontà - non voglio dire il coraggio - di archiviare tale indagine per mancanza totale di ogni indizio. Noi ci auguriamo

oggi o domani dopo un approfondimento - allo stato degli atti, non potendo comunque valutare l'interesse pubblico, dovremmo propendere, probabilmente, per una dichiarazione d'insussistenza dell'interesse pubblico e, quindi, autorizzare la procedura. Cosa paradossale: non avendo gli elementi per valutare l'esistenza dell'interesse pubblico, noi dovremmo dare l'autorizzazione. Tuttavia, sarebbe paradossale anche la decisione contraria, cioè quella di non autorizzare, perché non autorizzeremmo il seguito della procedura senza avere valutato l'interesse pubblico che poi, magari, da un'indagine più approfondita, potrebbe risultare insussistente. parlamentari ha fatto la sua scelta - e riprendo quanto ho detto all'inizio - non per lavarsi le mani da una decisione, ma per invitare il tribunale dei Ministri ad assumersi le sue responsabilità investire - eventualità che intuitivamente riteniamo non possibile allo stato degli atti, anche perché si tratta di una procedura più che datata

nei confronti di quest'Assemblea, ha la responsabilità di promuovere azioni che certamente, anche sul piano della notorietà e della pubblicità,

pur essendo la Giunta stessa in imbarazzo di fronte a quanto ci è stato trasmesso, poiché il caso era di tale palese infondatezza, nei confronti del professor Marzano, all'epoca

la legge prevede su questo genere di fattispecie. In particolare, il Ministro sarebbe stato ritenuto responsabile di

Il principale addebito che gli è stato avanzato è che una delle persone nominate era troppo giovane.

A questo punto, assunte tali notizie, il fatto che fosse di giovane età costituiva addirittura un dato positivo in più, perché se nonostante la giovane età, era già particolarmente reputato in questo campo, vuol dire che ciò non era dovuto solo alla lunga esperienza, ma evidentemente ad una particolare rapidità nell'apprendere e nell'esercitare in questo settore.

potuto trovare un lavoro perché meno qualificata o perché in età meno appetibile per eventuali futuri datori di lavoro. Per cui, l'azienda si trova di fronte a gravi difficoltà, se non a volte all'impossibilità ad andare avanti.

la manodopera, si trova ad essere completamente inutilizzato. Nel caso degli impianti è un peccato, perché è uno spreco per la collettività, ma nel caso delle maestranze è un grave problema sociale,

di questi amministratori, non soltanto che essi siano competenti, esperti e che non facciano errori né di procedura, né di amministrazione, ma che agiscano in fretta, altrimenti, pur praticando la migliore delle amministrazioni, pur compiendo i passi

perché nessuna norma, nessuna legge, nessun documento e nessun regolamento interno stabilisce i criteri sulla base dei quali il Ministro deve nominare gli amministratori. Si tratta di una discrezionalità che viene concessa in questo caso al Ministro, che può essere

L'autorevole senatore Biondi ricorda che anche i Sottosegretari sono nominati con criteri di discrezionalità, per cui addebitare al Ministro qualsivoglia

per dare contezza del nostro comportamento e soprattutto della decisione che è stata assunta e che alcune perplessità ha sollevato nelle parole del senatore Caruso. Ricordo anzitutto come la nostra richiesta come Giunta sia relativa all'applicazione delle previsioni dell'articolo 96 della Costituzione, che ha presupposti e requisiti molto particolari, anche per quanto riguarda le leggi costituzionali, poi attuative di questi princìpi, e non sia assolutamente una norma che possa farsi coincidere con l'impostazione dell'articolo 68 della Costituzione. La richiesta della Giunta, che è stata presentata in maniera dettagliata, soprattutto per quanto riguarda la parte di fatto

è una richiesta che viene presentata in Senato dopo una serie di approfondimenti, audizioni, acquisizioni documentali effettuate da tutti i membri della Giunta con estrema serietà. ci siamo trovati di fronte ad una situazione molto singolare perché l'autorità giudiziaria in quella sede ha affermato di trovarsi in presenza di elementi estremamente labili

proprio sulla base delle norme costituzionali e di tutta una serie di sentenze, anche recentissime, emanate dalla Corte costituzionale. La Giunta, dopo un'approfondita valutazione in fatto e in diritto, ha considerato tutti gli aspetti segnalati dal senatore Caruso, valutandoli anche nella delicatezza delle situazioni, ed è pervenuta ad una decisione unanime proprio perché in questa situazione di fatto e di diritto non si può decidere in maniera diversa. Si tratta di rispettare le norme costituzionali.

Terza ipotesi: se l'autorità giudiziaria decidesse di non esser d'accordo con la nostra impostazione, potrebbe sollevare il conflitto e sarebbe quindi la Corte costituzionale a valutare

Presidente, non so se il caso possa ritenersi infondato, comunque non abbiamo il diritto di intervenire nel merito. Credo che la proposta presentata dal relatore sia corretta perché rispetta in modo molto rigoroso il dettato costituzionale. Probabilmente, se il tribunale dei Ministri si fosse comportato diversamente all'inizio non ci troveremmo in questa situazione

non significhi perdere tempo e che sia nostro dovere agire in questa direzione. La normativa recata dalla legge costituzionale affida al tribunale dei Ministri il potere-dovere di delineare in modo preciso e puntuale le fattispecie dei reati sulla base di riscontri indagativi ampi e completi. Solo l'assolvimento di tale funzione permette alla Giunta e poi all'Assemblea di esprimere un giudizio circostanziato e lineare, sulla base - ripeto - del lavoro che deve essere svolto dal tribunale In questo caso il lavoro non è stato svolto secondo le condizioni che si dicevano prima: noi saremmo nella condizione di operare

al tribunale dei Ministri di valutare se si è davvero in presenza di un'ipotesi accusatoria, dotata di un ragionevole margine di fondamento,

in realtà siamo in presenza di una vicenda apparentemente molto complicata, di grande delicatezza, sulla quale le decisioni unanimi, se non ricordo male, della Giunta delle elezioni e delle immunità, questa specifica motivazione: una attenzione estrema a cosa il Senato deve deliberare in questa materia. Quando siamo chiamati ancora in sede di autorizzazione a procedere, istituto caducato anni fa come norma costituzionale e rivisto sotto vesti nuove in tema di responsabilità ministeriale, ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale gli elementi che ci vengono dati, a prescindere dalla nostra valutazione dei fatti, non sono tali da consentire un giudizio definitivo. Ecco perché, tra le ipotesi della Giunta, nessuna indica una qualunque valutazione sui fatti, ma ci limitiamo sostanzialmente a constatare che non abbiamo elementi sufficienti per poter deliberare. Mi sembra che il Senato debba tener conto del fatto che l'unanimità della Giunta è una manifestazione di volontà non di tipo partigiano; è una valutazione di ordine costituzionale molto serio e, per quanto mi riguarda, come componente della Giunta, ritengo, non come posizione personale, ma politica, di essere favorevole alle richieste del collega Manzione, soprattutto, in particolare, con riferimento all'intervento del collega Casson.

È meglio che sia singolare che plurale. Se il cittadino Marzano e gli altri fossero cittadini semplici, forse questa vicenda avrebbe avuto un corso diverso, più rapido, più coerente con le posizioni ricordate autorevolmente dal relatore e riprese da altri colleghi, in particolare dal senatore Casson, che ha fatto presente quali sono i vincoli in cui ci troviamo e che purtroppo - sto per dire - preterintenzionalmente, dal nostro punto di vista, si riverberano con la richiesta al giudice di essere tale: *iudex esto*, sii giudice! Invece non è avvenuto che il giudice abbia fatto quello che doveva fare sulla base degli elementi ricordati, di cui la Giunta si è fatta carico in termini di valutazione, di approfondimento e quindi di capacità di giudicare, sulla base di elementi che essa stessa ha considerato come non consistenti. Tuttavia, il paradosso vuole che di fronte a quello che il cittadino avrebbe dovuto avere dal giudice naturale precostituito per legge, non quello artificiale (la procura di Potenza che decide, nella sua potenza, di essere *erga omnes*), una decisione conforme ai diritti ed alle considerazioni che su questi stessi diritti i giudici responsabilmente sono chiamati a fare Invece, non è così! Oggi noi dobbiamo rimpallare al tribunale dei Ministri, per le ragioni costituzionali che sono state poco fa espresse e che sono giuste, una decisione che avvolge ancora nel sospetto il cittadino Marzano, ministro *pro tempore*. Questo, credo, sia un aspetto che ci deve far riflettere. Ieri ho ascoltato la requisitoria del senatore D'Ambrosio.

in relazione all'interesse che qualcuno ripone - tenuto conto della notorietà dei soggetti - di farsi, con lo specchio delle sue brame, la più bella del reame, nell'individuazione dei ruoli che ci si assegna a seconda della notorietà. Questo è uno dei casi. Siamo di fronte alla violazione di un brocardo latino

risposto all'esigenza di salvaguardare ciò che costituiva non una violazione, ma magari un errore, non dovuto, però, ad interessi patrimoniali, bensì all'esercizio di una facoltà che è garantita solo dalla libertà di valutazione della scelta nella discrezionalità e alle necessità poco fa esposte di provvedere,

Ministro della Repubblica da una responsabilità che non gli apparteneva? Lo sapremo alla prossima puntata, quando il tribunale dei Ministri

quando sarà investito dal giudice di un potere proprio che la Costituzione gli assegna). Mi permetto, allora, di dire che, se vi è una prova che tante questioni che attengono al rapporto tra il cittadino e la magistratura non possono essere risolte nelle tavole rotonde, ma devono essere affrontate in termini di effettiva relazione tra il diritto del singolo e il potere più alto dello Stato di dare giustizia quand'è necessario, forse davvero quest'Assemblea potrebbe essere una tavola rotonda, finalmente, per metterci d'accordo, non allontanarci dai problemi, non commissariare le decisioni, non sospendere gli esiti, non scoprire le tombe e far risorgere i morti, come una legge dello Stato che si fa

che per chi è laureato in legge è anche una mesta considerazione - che sono passati i tempi, ma ad avere ragione spesso si corrono maggiori rischi di quando si ha torto.

Signor Presidente, ho l'impressione che la proposta del collega Caruso non sia stata utilmente intesa. Il collega Caruso, anziché formalizzare formalmente una proposta all'Aula alternativa a quella riconducibile alla relazione svolta dal relatore sulla base della decisione assunta dalla Giunta (con il permesso dei colleghi), ha svolto invece una riflessione ad alta voce per indurre un ragionamento che, per altri versi, è stato proficuo, se è vero che le considerazioni che il collega Caruso ha rappresentato all'Aula sono state riprese da tutti gli altri colleghi, da Casson a Biondi, a Pastore, a Ripamonti, a Malan. Alla fine, collega Caruso, la considerazione che deve essere dirimente, rispetto alla scelta che quest'Aula andrà ad assumere fra poco, è che proprio nel rispetto della Carta costituzionale, che opera una delimitazione funzionale, riservando alla Giunta (quindi all'Aula e al Parlamento) solamente un apprezzamento sulle scriminanti speciali, dobbiamo comprendere come non esiste la possibilità di una valutazione di merito piena. Condivido quanto diceva il collega Biondi: ci troviamo al cospetto di una fattispecie che, nel merito, ci rappresenta una situazione all'interno della quale lo stesso Collegio per i reati ministeriali riconosce che non ci sono gli elementi per sostenere un'accusa e, nello stesso tempo, rimette una valutazione, chiedendo l'autorizzazione al Senato.

surrogare al Collegio per i reati ministeriali; ci porta, correttamente, a dire soltanto che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, per esercitare correttamente quel potere che la Carta costituzionale ci attribuisce, dobbiamo pretendere che detto Collegio emetta una valutazione che sia comprensiva di tutti i limiti che la legge gli attribuisce, di quei confini ampi, e non assuma invece l'atteggiamento di chi dice che da una parte certamente non c'è nessun rapporto fra l'ex ministro Marzano e coloro che sono stati nominati commissari, che certamente esiste una discrezionalità, ma che astrattamente è partito questo impulso. Non significa assolutamente niente.

sperando di aver riassunto in maniera corretta i limiti della proposta che il collega Caruso aveva fatto all'Aula. Tale proposta, se così fosse, sarebbe assorbita dalla proposta che invece formalmente ho rappresentato all'Aula. Signor Presidente, il relatore ha inteso correttamente; spero di non essere stato io ad esprimermi in maniera tanto incerta da creare confusione e far malintendere a lei, signor Presidente, e alla Presidenza in definitiva. Ho esordito nel mio intervento

Ho fatto questo non per banale piaggeria, né nei confronti del relatore, né nei confronti della Giunta stessa; ma per introdurre un ragionamento che ha poi portato, come conclusione - speravo di averlo detto chiaramente, ma evidentemente così non è stato non ad una proposta alternativa all'Aula, su cui sarebbe stato quindi necessario esprimere un voto, ma ad una proposta al relatore di riconsiderare la questione, per egli proporre, ove vi fosse stata una prognosi favorevole nella riconsiderazione, che l'affare riguardante il professor Marzano ritornasse alla Giunta, per essere riconsiderato affinché la proposta della Giunta proposta della Giunta all'Aula fosse quella dell'archiviazione. Conosco bene i limiti della Giunta, signor Presidente. Se si vuole intendere il mio intervento anche con un contenuto minimamente provocatorio lo si può certamente fare. Esso era da intendersi nel senso che nel bilanciamento degli interessi costituzionali protetti, forse la Giunta avrebbe potuto concludere, a fronte della manifesta infondatezza delle accuse nei confronti del professor Marzano, riconosciute dal Collegio per i reati ministeriali, per la manifesta infondatezza della domanda proposta dal

Signor Presidente, intervengo brevemente per rappresentare all'Aula, nonché alla Presidenza innanzitutto, una vicenda che non può non interessare il Senato. Come tutti sanno la Commissione giustizia, presieduta dal senatore Salvi, ha disposto un'indagine conoscitiva su tutte le questioni attinenti alle intercettazioni telefoniche, indagine conoscitiva che abbiamo utilmente portato avanti nei mesi di luglio e settembre e che abbiamo ultimato, se non fosse per una coda che dovrà essere completata nella nella prossima settimana. Il dato che mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea è collegato all'ordinanza di custodia cautelare

con una serie di audizioni a tutto tondo che ci hanno portato, ad esempio, ad ascoltare il professor Franco Pizzetti, presidente dell'*Authority* il quale, giustamente, ci indicava quale fosse l'alveo all'interno del quale, per cercare di regolamentare al meglio le intercettazioni telefoniche, dovessimo muoverci. Egli lo individuava da un lato nel sistema relativo alla giustizia - mi riferisco agli operatori

garantissero un patrimonio comune assolutamente indiscutibile, che attiene alla massima garanzia di riservatezza rispetto ad alcuni dati sensibili e personali che non possono in alcun modo essere violati. Ciò che Ciò che accade a Milano, signor Presidente, ci lascia comprendere come non si deve soltanto ragionare di un alveo all'interno del quale

di monopolio obbligato. Voglio dire che nel momento in cui la magistratura chiede che vengano svolte delle intercettazioni telefoniche e chiede queste, che vengono definite in gergo prestazioni obbligatorie, non può scegliere il gestore. È evidente infatti che se chiede di sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica del senatore Manzione sarà la scelta compiuta a monte dal senatore rispetto al gestore che determinerà chi sarà tenuto ad eseguire la prestazione obbligatoria. sappiamo che questo è un meccanismo che non è possibile pretendere venga controllato direttamente dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, signor Presidente, abbiamo riscontrato che il massimo dei gestori, e mi riferisco al gruppo Telecom, cioè quello che proprio perché si tratta di prestazioni obbligatorie rende il maggior numero di tali prestazioni sia per quanto riguarda la rete fissa che quella mobile, è un gruppo che - sulla base delle cose che abbiamo appreso e mi sembrano inconfutabili, poi dirò perché conduce delle indagini parallele, gestisce degli archivi alternativi, esercita una forma di intercettazione rispetto a tutti gli utenti perché rappresenta un colosso in questo settore. riscontrata tale situazione - e mi rivolgo anche al presidente della 2a Commissione, il collega Salvi - porci soltanto il problema di ragionare di come garantire la riservatezza e la segretezza di queste intercettazioni telefoniche senza preoccuparci del fatto che il massimo, il più grande dei gestori, anziché limitarsi ad eseguire queste prestazioni obbligatorie che gli vengono richieste dalla magistratura, si preoccupa invece di determinare indagini parallele, archivi informatici e una serie di operazioni che vengono definite dal «Corriere della Sera», uno dei tanti giornali che abbiamo potuto leggere stamattina, come

fare questo intervento sull'ordine dei lavori approfittando del fatto che dovendo subito dopo riprendere la discussione generale sulla proposta di modifica, o meglio di sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, è presente in Aula il rappresentante del Ministero della giustizia. È un rappresentante qualificato; non abbiamo il ministro, il senatore Mastella, che di solito quando si svolgono le discussioni generali non c'è mai, ma abbiamo comunque la presenza di un rappresentante qualificatissimo del Ministero della giustizia. Voglio chiedere proprio al Ministro della giustizia se non sia il caso di cominciare a valutare come proprio queste prestazioni obbligatorie, che obbligatoriamente vengono chieste a quel gestore telefonico, non offrono più garanzia. È inutile che ragioniamo delle regole, di come vengono gestiti gli archivi o di come le notizie riservate che entrano a far parte del materiale processuale devono essere gestite, quando a monte l'affidabilità del gestore principale non c'è più. Vorrei allora allora che la Presidenza si facesse carico di chiedere al Ministro della giustizia di venire in Aula a discutere su questa delicatissima questione, anche per rappresentare al Senato se non sia opportuno in questa condizione, dopo avere sentito l'autorità garante, valutare anche la possibilità di chiedere una sospensione della concessione che per il momento è stata rilasciata alla Telecom - proprio rispetto a quelle prestazioni obbligatorie che non sono più assolutamente garantite. È chiaro che questo è un invito che rivolgo anche al presidente Salvi perché, all'interno di quel circuito di audizioni che abbiamo messo in campo, un avvenimento come questo che ha diretta rilevanza non può assolutamente essere trascurato.

Presidente, non posso nascondere a me stesso e non esprimere le preoccupazioni che abbiamo tutti quando vengono fuori queste vicende. Non voglio entrare nel merito delle problematiche sollevate dal collega Manzione se non per quanto riguarda i lavori

con la Commissione affari costituzionali. Perché dico questo? Ricordo brevemente, Presidente, ciò che è accaduto in questi mesi dall'inizio della legislatura. Il tema delle intercettazioni è stato assegnato alla Commissione giustizia, che ha iniziato anche un'indagine conoscitiva ritenendo, proprio come diceva il senatore Manzione, che il tema interessasse, sostanzialmente,

cioè che il tema dell'uso o dell'abuso delle intercettazioni non si limitasse al segmento strettamente giudiziario della ricerca e della scoperta

recenti e quantomeno al sospetto, se non alla prova, che in realtà si sia creata un'organizzazione più o meno strutturata che intercetta le comunicazioni e utilizza i tabulati e le conversazioni di cittadini privati, più o meno autorevoli e più o meno noti, per una sorta di mercato globale della riservatezza, credo che la

di chi ha in questa materia una competenza anche formale. Pertanto, esaurita l'indagine conoscitiva della Commissione giustizia, è a mio parere necessario procedere ad un intervento legislativo che non si limiti e non si fermi al corno del dilemma di cui parlava Manzione ma che investa tutto questo delicatissimo settore. Credo che ciò sia fondamentale e mi auguro che in tale occasione la Presidenza abbia la sensibilità di riconoscere a entrambe le Commissioni il ruolo e le funzioni che a loro competono su questo tema assolutamente fondamentale. [BRUTTI

con riferimento al raccordo tra pubblici ufficiali infedeli, che compiono attività illegittime, e strutture o persone all'interno della Telecom, che collaborano o abbiano collaborato ad attività illegittime. La terza componente è rappresentata da attività, anch'esse contro le leggi, che vengono svolte da agenzie investigative private. Il Parlamento ha certamente un potere di controllo su questa materia, poiché essa riguarda dati sensibili rientranti nella sfera privata di persone, esponenti istituzionali, uomini politici uomini politici e poiché sono in discussione attività illegittime compiute da pubblici ufficiali. Tale potere di controllo non può che essere svolto dall'organo parlamentare, il quale da un lato dà maggiori garanzie, per la riservatezza che circonda o dovrebbe circondare i suoi lavori, i suoi lavori, e dall'altro è abilitato a trattare dati sensibili e documenti riservati. Mi riferisco al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza, presieduto - come è noto - da un parlamentare dell'opposizione,

al di là dell'accertamento delle responsabilità penali, debba essere sottoposta al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza. Inoltre, credo che la Commissione giustizia debba concludere al più presto la propria indagine conoscitiva e inviarne le conclusioni inviarne le conclusioni all'Aula, in modo tale che su quei testi, su quei resoconti, sulle acquisizioni di quella Commissione si possa svolgere una discussione, che può essere utile all'Aula e al lavoro che a mio avviso essere avviato in Commissione affari costituzionali, ai fini della determinazione di una disciplina nelle materie che noi riteniamo malamente disciplinate. questo momento ciò riguardi il Ministro della giustizia, quindi non mi pare sia necessario o utile in questo momento una discussione con il sottosegretario Scotti o il Ministro della giustizia. Ritengo che dobbiamo mettere sui binari che ho indicato il lavoro da svolgere, sapendo che ci troviamo di fronte ad una serie di gravi abusi e che si deve intervenire in questo campo con senso di responsabilità, con la consapevolezza che abbiamo a che fare con un'azienda quotata in Borsa, ma anche con la fermezza e la decisione di andare fino in fondo nello scoprire e nel sanzionare gli abusi che incidono sulla vita della democrazia italiana.

emersero fatti che poi si sono rivelati in maniera clamorosa in queste giornate. Nel corso dell'audizione di funzionari Telecom, questi risposero alle domande dei commissari e dovettero ammettere - ho buona memoria che alcune patologie stavano attraversando la vita della società e avevano dato luogo ad iniziative giudiziarie, la cui portata all'epoca non era nota come lo è oggi. Condivido la preoccupazione, signor Presidente, che ha manifestato il collega Manzione e che poi gli altri colleghi intervenuti hanno rimarcato. Ritengo che il luogo deputato a trattare in maniera maniera più approfondita queste vicende debba essere sia la Commissione che il Comitato di controllo sui servizi, viste le connessioni perverse di cui oggi abbiamo letto sui giornali e che ci lasciano stupiti,

vede, Presidente, la coincidenza fra le questioni complesse che stanno attraversando la realtà finanziaria, gli assetti proprietari e patrimoniali di Telecom

cosa sia accaduto e cosa stia accadendo nell'ambito di tale gigante dell'economia, che impegna 80.000 uomini (il mondo del lavoro è fortemente preoccupato per quanto accade). Soltanto oggi sembra che si sia scoperto come siano avvenuti, nel corso di questi anni, alcuni ineffabili passaggi di proprietà (signor Presidente, gente senza denaro ha comprato Telecom!): tutte queste realtà così particolari meritano una risposta. Vi sono due momenti apparentemente sconnessi fra loro, ma intimamente connessi. Da una parte, irrompe l'autorità giudiziaria, rilevando la sussistenza di un'associazione a delinquere che utilizzava gli strumenti e le alte tecnologie che la società ha a disposizione per spiare parlamentari, imprenditori, cittadini comuni. E che fine hanno fatto

allora, che una vicenda così grave, proprio in concomitanza con l'iniziativa giudiziaria cui benemeritamente ha fatto cenno il collega Manzione, imponga

che venga il Presidente del Consiglio a rispondere anche su tali tematiche che certamente non sono secondarie nel contesto che riguarda Telecom.

Sono state sollevate questioni di grande peso e rilievo, e si è parlato anche dell'attività in corso da parte della Commissione giustizia, che ho l'onore di presiedere: ritengo, pertanto, opportuno e necessario spendere qualche parola sull'argomento. Effettivamente - secondo quanto ha ricordato il senatore Manzione, come i colleghi della Commissione giustizia presenti in Aula potranno testimoniare - l'indagine conoscitiva da noi avviata, ormai prossima alla conclusione, aveva già fatto emergere, nei limiti, naturalmente, della strumentazione di cui il Parlamento dispone, il caso che oggi è esploso sulla stampa. In primo luogo, è emersa un'estrema vulnerabilità dei sistemi utilizzati ai fini delle intercettazioni telefoniche. Proprio la modernità degli strumenti attualmente attualmente usati non dà sufficienti garanzie che le intercettazioni legittime rimangano nel novero dei soggetti alle quali sono destinate, pertanto la caccia che consuetudinariamente si fa quando escono notizie sui giornali a delimitate categorie - magistratura, Polizia di Stato e, da una certa fase in poi, avvocatura - probabilmente, anzi certamente, va estesa.

visto che si discute tanto dei costi delle intercettazioni. Mi domando se debbano essere posti a carico dello Stato e non di quei soggetti che, essendo titolari di concessioni, ne ricavano altri e cospicui guadagni. Questo aspetto ha un certo rilievo, ma non è il punto che è stato sollevato.

l'iniziativa della Commissione giustizia possa proseguire, se i colleghi della Commissione concorderanno, nell'ufficio di Presidenza, con queste due audizioni, dopo le quali saremo pronti per riferire. Il Governo,

c'è da approfondire l'iniziativa legislativa, lo faccia la Camera dei deputati, su sollecitazione del Governo, tenendo conto però che i temi emersi in questa materia al novanta per cento non sono affrontati dal disegno di legge del Governo che si occupa, invece, di altre questioni pur rilevanti: della tutela della *privacy*, della riservatezza e così via.

è vero che la Commissione terminerà il proprio lavoro, con riferimento all'indagine conoscitiva, attraverso un documento e la proposizione all'Aula delle conclusioni cui essa sarà pervenuta. è intuitivo, logico e razionale anche il fatto che, su questo tema, al di là del documento scritto, i singoli componenti della Commissione hanno acquisito conoscenze, sensibilità e opinioni che, fisiologicamente, travalicano lo scritto. Quindi, non ha senso Quindi, non ha senso la scelta che è stata operata - che poi sappiamo essere, a volte, una scelta non consapevole, figlia della burocrazia più che della determinazione - dell'affidamento all'altro ramo del Parlamento del disegno di legge del Governo su una materia che, a mio modo di vedere, trattata complessivamente, se possibile, in tutti i suoi aspetti, attraverso una disciplina quadro. Ebbene, non è razionale che questo disegno di legge sia affidato all'altro ramo del Parlamento. A ciò vi sono rimedi: sia il Regolamento del Senato che quello della Camera dei deputati riportano tale questione e ne disciplinano il rimedio. Le chiedo, signor Presidente, di voler avviare le due soluzioni possibili: la prima, nei confronti del Ministro per i rapporti con il Parlamento, affinché sia il Governo a riconsiderare l'opportunità di affidare a questo ramo del Parlamento e non all'altro

con grande garbo e nettezza dal senatore Valentino, sono già state esposte a chi oggi verrà a riferire il parere del Governo sulla vicenda Telecom. Sono già state affrontate in un'altra fase; quindi, su queste non ho da aggiungere altro.

di cui ovviamente ho apprezzato l'intervento - come anche gli altri - che oggi pomeriggio, alle ore 14,30, la Commissione affari costituzionali deciderà sulla proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra la libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica, che è un elemento connesso, se non proprio centrato su questo aspetto, che riguarda più generalmente i temi in discussione.

che, da Camera alta, noi si sia diventati «anti-Camera». Neppure il Ministro della giustizia oggi è qui ad ascoltare la discussione sulla modifica dell'ordinamento giudiziario; inoltre, siamo privati della presenza ormai

dopo oltre cinquant'anni di attesa di riforma per l'ordinamento giudiziario, finalmente con la legge n. 150 del 2005 l'*iter* si è concluso. Com'era prevedibile, sotto la pressione dell'Associazione nazionale magistrati, il Governo, non per migliorare la legge ma con l'intento di cancellarla definitivamente, ha presentato l'Atto Senato n. 635, a firma del ministro Mastella, che, in un solo colpo, vuole sospendere l'efficacia dei decreti nn. 106 del 20 febbraio 2006, 109 del 23 febbraio 2006 e 160 del 5 aprile 2006. Se dovesse essere approvata, la presente proposta sarebbe senza dubbio una vittoria della ANM sul Parlamento, un *vulnus* inaccettabile per la democrazia. È evidente che il ministro Mastella, con il sostegno della ANM, vuole cancellare completamente la riforma Castelli, unico atto legislativo che ha portato riforme fondamentali nel campo della giustizia. Mi corre l'obbligo ricordare che, dopo una riflessione approfondita, nella quale in più riprese successive il ministro della giustizia Castelli è venuto sempre più incontro alle richieste sia della magistratura, delle forza politiche (anche dell'opposizione), desta sconcerto riscontrare come ancora oggi si parli di questa come una riforma ingiusta, che aggrava l'inefficienza della giustizia italiana ed attenta all'indipendenza e all'autonomia di tutti i magistrati. Al contrario, noi riteniamo che questa riforma rappresenti un'innovazione fondamentale in materia di giustizia, dato che, per la prima volta da oltre cinquant'anni, viene modificata la legge fondamentale in materia di ordinamento giudiziario, risalente al lontano 30 gennaio 1941. Si tratta di una riforma che incide sull'organizzazione interna della magistratura, tentando di ridisegnare il sistema di accesso in magistratura in modo tale da recuperarne la professionalità, l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità. In sostanza viene a delinearsi un sistema più puntuale nella valutazione dei magistrati. A tal fine, per essere ammessi al concorso, non basta più la semplice laurea in giurisprudenza, ma sono richiesti ulteriori titoli abilitanti; dovranno essere sostenuti colloqui di idoneità psicoattitudinale volti a valutare la predisposizione del candidato, anche in riferimento alle specifiche funzioni che egli avrà indicato al momento della domanda di ammissione al concorso; si dovrà seguire un apposito corso di formazione iniziale presso la scuola della magistratura e di seguito trascorrere i periodi dell'uditorato presso i vari uffici giudicanti, requirenti e di prima assegnazione, così che il periodo di tirocinio iniziale serva per valorizzare la formazione dell'uditore attraverso l'apporto di varie esperienze diverse. Grazie a questa riforma, finalmente anche la progressione in carriera dovrà svolgersi alla luce di profili meritocratici, venendo sganciata dal semplice avanzamento per anzianità di servizio ed affidata a momenti di effettiva valutazione (concorsi) oltre che a corsi di aggiornamento professionale. In pratica, queste innovazioni cambiano la prospettiva dalla quale si deve guardare al superamento del concorso: l'essere diventati magistrati non significa più aver raggiunto un traguardo nella vita, ma un semplice punto di partenza verso una funzione che richiede costantemente impegno professionale ed aggiornamento continuo, perchè il magistrato aggiornato è anche più qualificato dal punto di vista professionale. È utile ricordare che il decreto legislativo n. 106 del 2006 recava: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (...)», cioè la ristrutturazione

nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati (...)». L'intento del presente disegno di legge è di sospendere l'efficacia dei sopra nominati decreti al 31 luglio 2007 ma, in realtà, il vero scopo è di sospenderli per sempre. Se questo provvedimento venisse approvato, signor Presidente, il nostro Paese diventerebbe l'unica democrazia al mondo in cui l'organismo legislativo (quindi il Parlamento) deve sottostare al ricatto dell'organismo che applica le leggi (quindi la magistratura): un bel colpo mortale alla legalità e alle istituzioni democratiche. Questa proposta non è intenzionata, come sostiene il Ministro, a migliorare alcuni aspetti della riforma Castelli. Il vero obiettivo è quello di accontentare la potente casta delle toghe, che da cinque anni non fa altro che criticare ciò che il Parlamento approva. Signor Presidente, con il presente atto non si vuole modificare - cosa peraltro legittima - una legge attualmente in vigore,

mi dispiace che non sia presente in Aula - non ha citato alcun effetto negativo della legge n. 150 del 2005 perché, evidentemente, il Ministro non ne ha rilevati e non voleva essere questo lo scopo dell'intervento. L'intenzione

Se la presente proposta venisse approvata sarebbe sancita la definitiva abdicazione del potere politico di fronte alla magistratura. La giustizia sarebbe governata esclusivamente dal volere e dalle proposte dei magistrati. Questo provvedimento è l'inizio dell'azione legislativa del presente Governo di sinistra, il cui motto è: cancellare tutto quanto fatto dal precedente Governo. Il Parlamento non può rinunciare al suo ruolo sancito dalla Costituzione, che la sinistra cita sempre come intoccabile, e non può subire il ricatto da parte di alcuno. Voglio, infine, ribadire che l'approvazione della presente proposta sancirebbe l'abdicazione dell'istituzione democratica di fronte a una magistratura sempre più decisa a condizionare il Parlamento ed il Governo con le proprie volontà

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, signori rappresentanti del Governo, intervengo quasi al termine della discussione generale di un disegno di legge specialissimo, quale è questo, che non mira a realizzare alcuna positiva proposta legislativa, ma che intende sospendere l'efficacia, futura, di tre leggi già in vigore da qualche mese, attuatrici di alcune (e significative) parti della riforma dell'ordinamento giudiziario, riforma che il Governo di centro-destra riuscì a realizzare, dopo ben sessant'anni dalla norma costituzionale che la prescriveva e dopo gli innumerevoli insuccessi collezionati sul punto, nel corso del tempo, da vari Governi e dalle più assortite maggioranze. Più qualche altra cosa, di non trascurabile rilievo, su cui sarà anche bene spendere qualche parola nel corso del dibattito. Intervengo a ridosso del momento in cui il Ministro della giustizia ha finalmente inteso spiegare al Parlamento quanto il Parlamento stesso (trasversalmente, nelle sue componenti di maggioranza e di opposizione, anche attraverso voci istituzionalmente e politicamente autorevoli - penso al presidente Salvi) gli aveva chiesto di spiegare fin dal momento in cui questo disegno di legge si fece strada fra i lavori del Senato. E cioè, quali parti egli in realtà non condividesse delle tre leggi di cui proponeva di sospendere l'efficacia. Quali parti, delle tre leggi, badate bene, colleghi (e non le leggi nel loro complesso), perché diversamente di altro avremmo parlato e ben più radicale avrebbe dovuto ragionevolmente essere la proposta legislativa del Ministro, nel senso dell'abrogazione *tout court* (pura e semplice) delle ripetute tre leggi: soluzione radicale (e, come detto, assai semplice), certamente gradita alla categoria professionale che in tutta evidenza assiste, circonda e controlla, forse tiene prigioniero l'attuale Ministro, ma forse troppo ardita e coraggiosa per un Ministro (come l'attuale), che è anche uomo politico troppo avvertito, intelligente e raffinato, per non sapere, che una simile scelta sarebbe stata, sì, gradita all'agguerrita e potente truppa dei 9.000 magistrati, ma anche viceversa assolutamente invisa ai 150.000 avvocati, per esempio, che peraltro già ora sono in sciopero - come noi tutti sappiamo - per distinta ragione, e per fatto di altro Ministro di questo Governo. E non solo. secondo luogo, del pari di quella - recente - dell'indulto, sarebbe stata ben difficilmente compresa e comprensibile per i cittadini che, attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, avevano appena conosciuto - questo ci rimanda a quanto discusso non più di mezz'ora fa parlando della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del professor Marzano

(in maniera equa, ma soprattutto seria e finalmente effettiva, e finalmente «obbligatoria», tutte le volte in cui nella condotta da lui tenuta, nei confronti del cittadino stesso (o della collettività di essi), fosse stata ravvisata scorrettezza, o lesività di diritti, o fosse anche stata semplicemente superata la soglia dell'al di là delle righe o della contrarietà ai doveri. Un intervento, quello di ieri l'altro del Ministro, dunque assai atteso e assai importante, perché attraverso lo stesso sarebbe stato finalmente possibile, soprattutto per l'opposizione, sciogliere un serio dubbio che è fin qui aleggiato; sarebbe stato, cioè, possibile capire se la proposta di sospensione avanzata dal Governo costituiva presupposto concreto di una proposizione seria, migliorativa della riforma dell'ordinamento giudiziario, oppure se si trattava soltanto di una cambiale firmata in campagna elettorale dall'attuale maggioranza e che a lui, Ministro, toccava ora di pagare. Il dubbio - come detto - era aleggiato ed anche da me era stato personalmente manifestato, durante i lavori in Commissione giustizia. Ma in quella fase il Ministro aveva più volte ripetuto che egli non intendeva «blindare» nulla (come in gergo, e me ne scuso, ci si è abituati a dire), che egli offriva e attendeva dialogo con tutte le parti politiche e che occorreva lavorare insieme, nell'interesse dello Stato, nell'interesse della giustizia e così via (insomma, un po' quanto ancora ha ripetuto l'altro ieri, con un'impudenza - chiedo scusa, signor Presidente - degna di miglior causa). A fronte di ciò fu dunque obbligatorio che si facesse strada, rispetto al dubbio, il dovere istituzionale (che è anche un dovere dell'opposizione) di assegnare credito a chi è chiamato a svolgere la delicata funzione che è propria dell'unico Ministro cui la nostra Costituzione riserva esplicito ed espresso richiamo, a chi - senatore Mastella - è, da questo punto di vista (quello della presunzione di sincerità e del conseguente credito), il Ministro di tutti e non solo di una parte politica o di una parte parlamentare. E a fronte di ciò fu dunque stabilito, da parte delle forze di opposizione, che l'appropriata risposta dovesse essere quella del dibattito franco e leale, oltre che - positivamente quello della presentazione di pochi emendamenti, tra i quali pochissimi quelli, per così dire, di bandiera e tutti propositivi e migliorativi i rimanenti: così è stato e ciò corrisponde alla precisa manifestazione, durante i lavori coordinati dal presidente Salvi, della non volontà di praticare ostruzionismo alcuno e della decisione di dare viceversa credito al Ministro e alle sue affermazioni. La risposta alla risposta è del tutto nota: è del tutto nota: un solo emendamento approvato, del Governo, addirittura banalmente peggiorativo della proposizione iniziale. Il dubbio, onorevoli colleghi, non è stato più dubbio, ma è divenuto certezza: il disegno di legge di sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario era (è sempre stato e pacificamente è) il banale, modesto, non nobile pagamento di un debito politico della maggioranza di Governo, di una cambiale elettorale in favore di una *lobby* autorevole e potente, quale è quella dei magistrati. Il senatore Mastella ha accettato, quale «Ministro alla partita», di esserne l'ufficiale pagatore. Con personale tornaconto o senza è un problema che assolutamente non ci appassiona e non ci interessa. Sono e restano problemi del Ministro. Quello che ci interessa è, tuttavia, che il Ministro si è condotto, e si conduce, in questa vicenda in maniera evidentemente non sincera: non solo, alla luce delle reiterate (e non praticate) profferte di dialogo, ancora l'altro ieri declamate qui in Aula, ma, anche e soprattutto, in relazione al merito della questione che ben probabilmente non è invero quello della transitoria sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni, ma quello (peraltro praticato in maniera vile) del definitivo affossamento di una riforma che pure riguardava contesti di grande utilità per gli equilibri del Paese e per i suoi cittadini. Nulla vi è stato, nel nostro passato politico, di più definitivo del provvisorio e vedrete che anche questa volta così sarà. Se mi sarò sbagliato, signor Ministro, sarò lieto di dargliene atto, come lieto sarei stato per altra e gravissima questione che pure la riguarda molto, molto da vicino. Il ministro Mastella, signor Presidente, è quello stesso che - intervenendo in Commissione giustizia e qui nell'Aula del Senato e, ancora, davanti ai deputati, allora accompagnato dal suo sottosegretario Manconi non esitò a comunicare al Parlamento dati gravemente difformi dal vero su una questione, la cui straordinaria delicatezza non è dato di revocare in dubbio, e su cui il Parlamento doveva proprio in quel momento formare la propria definitiva e doveva responsabilmente formarla proprio anche sulla base di quei dati che il Ministro era tenuto a dare, possedendoli alla luce ed in forza delle sue prerogative. Mi riferisco, signor Presidente, alla questione dell'indulto, che è definitivamente superata dal punto di vista legislativo (chi ora interviene, signor Presidente, appartiene ad una comunità politica che le leggi tende ad osservarle e ad accettarle e non a sospenderle), ma che lascia - proprio dal punto di vista politico - lo strascico logico del problema che l'inveridicità delle comunicazioni del Governo al Parlamento determina. Sostenni nel corso di quel dibattito che, per effetto del provvedimento in procinto di essere approvato, sarebbero stati anzitempo liberati oltre ventimila detenuti, senza contare i benefici che avrebbero determinato l'assenza di ogni controllo di sicurezza su altre decine di migliaia di condannati. Venne più volte ribadito dal Ministro e dal sottosegretario Manconi, con grande sicumera, in Commissione e in Aula, oltre che comunicato (e conseguentemente pubblicato) da giornali e televisioni, che il numero stimato (fino, addirittura, all'indicazione dell'unità) dei detenuti di prossima liberazione era assolutamente inferiore a quanto da me indicato e puntualmente doveva essere valutato in esattamente 12.756 unità. Il Parlamento, signor Presidente, su quei dati forniti dal Governo (che pure lasciavano perplessa la parte evidentemente più avvertita dei colleghi della maggioranza) prese la sua finale decisione, e questa finale decisione fu quella della concessione di un indulto, con i limiti e le esclusioni stabilite, perché dalle stesse derivassero i numeri che il Ministro aveva comunicato. Il «Corriere della Sera» dello scorso venerdì 8 settembre (data spero singolarmente non casuale per il Governo di cui lei, Ministro, fa parte) racconta agli italiani che lei invece, di detenuti, non ne ha liberati 12.756, non ne ha liberati 12.756, ma ben 21.000: un migliaio in più di quanto io avevo sostenuto che sarebbe stato. Io, signor Presidente, ero stato prudente nel mio intervento, non avevo mentito e non mi ero sbagliato. Il Ministro e il sottosegretario Manconi, invece, o mentirono o semplicemente si sbagliarono. Ma quasi del doppio? Dovete essere voi, colleghi di maggioranza, prima di ogni altri, a formarvi le convinzioni e a trarre le conclusioni che preferite. Perché a voi, prima che ad ogni altri, i cittadini chiederanno il conto, e di dare conto. Se il Governo in quell'occasione sbagliò, lo fece - come detto - sottovalutando un fenomeno delicato praticamente del cento per cento. Se il Governo, il Ministro e il Sottosegretario invece mentirono, è pacifico che ci si trovi di fronte ad un *impasse* anche istituzionale non certo trascurabile. Sono un realista, signor Presidente, e so bene che il mio invito ai colleghi tale resterà. Ma una cosa tuttavia mi domando. Errore inescusabile o condotta disinvolta che sia stata in quell'occasione quella del ministro Mastella, si può fare ancora finta di nulla anche ora? Si può permettere che oggi il Ministro - su altra e delicata questione - ancora reiteri disinvolte condotte? Senatore Mastella, ho nella memoria quello che mi sembra l'unico precedente della storia repubblicana di mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Ministro (di un Ministro guardasigilli, per l'appunto). Ragioni di simpatia personale mi inducono ad augurarle che non capiti anche a lei di trovarsi ad assistere ad analoga discussione, ma prudenza forse vorrebbe che lei si dia una mano da sé, mutando la propria condotta: non solo nei confronti della sua opposizione, ma anche per la sua maggioranza, nelle cui file militano persone cui certamente non manca il senso dello Stato e delle istituzioni, che sanno quello che vogliono e che non accettano (e non intendono che per esse si accettino) non degne scorciatoie. Una soluzione c'è. Avvicendi urgentemente il sottosegretario Manconi, per la ragione che preferisce lei, signor Ministro: per aver mentito al Parlamento, per inadeguatezza, per averle fornito dati gravemente fuorvianti su una questione delicata e decisiva. Veda lei. E accetti che le leggi in vigore tali restino e presenti al più presto le sue concrete proposte. Che saranno immediatamente esaminate, senza pregiudizio e in quella effettiva logica di costruttiva collaborazione che già una volta l'opposizione ha dimostrato di sapere e di poter accettare. Si tratta, come lei stesso ancora ieri ci ha ripetuto, signor Ministro, di norme tutto sommato non innumerevoli e lei ha, a suo corredo, anche fior di altri collaboratori, tecnici e politici. Non si limiti a pagare le cambiali, e faccia quello che ha sempre fatto: politica seria, nell'interesse dello Stato. E anche lei, come la saggezza popolare usa dire da sempre («dagli amici mi guardi invochi la necessaria assistenza. C'è un suo compagno di coalizione, un suo collega Ministro, che, oggi, si fa leggere sul quotidiano «la Repubblica», informando i cittadini del fatto che, a fronte di chi fa sforzi per il miglioramento dell'economia e per tante altre cose, di Ministro «ce n'è uno contrario che mira a inciuciare, a mettersi d'accordo sulle piccole questioni (...), una politica degli amici per gli amici, per gli amici, tutta mirata a salvaguardare i propri interessi». È lo stesso suo compagno di coalizione, senatore Mastella, che dice che «sui valori della legalità non si va a spanne»

sia profondamente lamentato per il sistema giudiziario e per tutti i problemi ad esso collegati. Finalmente, nella scorsa legislatura, si riuscì a fare una riforma che potrebbe, se non affossata, portare a significativi miglioramenti nel mondo della giustizia. Dopo una riflessione approfondita, nella quale in più riprese successive il ministro della giustizia Castelli è venuto sempre più incontro alle richieste sia della magistratura che delle forze politiche (anche di opposizione) di allora, desta sconcerto riscontrare come ancora oggi si parli di questa come di una riforma ingiusta, che aggrava l'inefficienza della giustizia italiana ed attenta all'indipendenza e all'autonomia di tutti i magistrati. Al contrario, noi riteniamo che questa riforma rappresenti un innovazione fondamentale in materia di giustizia, dato che, per la prima volta da oltre cinquant'anni, viene modificata la legge fondamentale in materia di ordinamento giudiziario, risalente al lontano 30 gennaio 1941. Si tratta di una riforma che incide sull'organizzazione interna della magistratura, tentando di ridisegnare il sistema di accesso in magistratura in modo tale da recuperarne la professionalità, l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità. In sostanza viene a delinearsi un sistema più puntuale nella valutazione dei magistrati. A tal fine, per essere ammessi al concorso, non basta più la semplice laurea in giurisprudenza ma sono richiesti ulteriori titoli abilitanti; dovranno essere sostenuti dei colloqui di idoneità psico attitudinale volti a valutare la predisposizione del candidato, anche in riferimento alle specifiche funzioni che egli avrà indicato al momento della domanda di ammissione al concorso; si dovrà seguire un apposito corso di formazione iniziale presso la scuola della magistratura e di seguito trascorrere i periodi dell'uditorato presso i vari uffici giudicanti, requirenti e di prima assegnazione, così che il periodo di tirocinio iniziale serva per valorizzare la formazione dell'uditore attraverso l'apporto di varie esperienze diverse. Grazie a questa riforma, finalmente anche la progressione in carriera dovrà svolgersi alla luce di profili meritocratici, venendo sganciata dal semplice avanzamento per anzianità di servizio ed affidata a momenti di effettiva valutazione, (come i concorsi) oltre che a corsi di aggiornamento professionale. In pratica, queste innovazioni cambiano la prospettiva dalla quale si deve guardare al superamento del concorso: l'essere diventati magistrati non significa più aver raggiunto un traguardo nella vita, ma un semplice punto di partenza verso una funzione che richiede costantemente impegno professionale ed aggiornamento continuo, perché il magistrato aggiornato è anche il più qualificato dal punto di vista professionale. Ma la riforma è interessante anche perché vuole garantire il principio costituzionale di terzietà del giudice, in attuazione del principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione. A tale scopo delinea il quadro della separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri, onde porre fine ad una commistione inaccettabile tra chi sostiene l'accusa e chi giudica, con la possibilità, oltretutto, di passare tranquillamente da una funzione all'altra in un modo che giudichiamo, a dir poco, inquietante. È bene precisare che la riforma non sconvolge il sistema, ma prevede appunto un meccanismo che si può definire di separazione, tendenziale e di fatto, delle funzioni: pubblici ministeri e giudici continuano, entrambi, ad appartenere all'ordine giudiziario, con la differenza che, attraverso la riforma, il passaggio dalle une alle altre funzioni viene subordinato ad una serie di condizioni che si presentano come sbarramento alla continua commistione tra le stesse cui abbiamo assistito fino ad oggi. Sotto questo profilo sono stati ripetuti gli attacchi da parte del mondo della magistratura, che lamenta un vero e proprio attentato alla sua indipendenza ed autonomia. In effetti, questa critica sembra dimenticare completamente quanto sia necessario distinguere le due funzioni, in ragione della diversa professionalità che l'esercizio delle stesse presuppone. Al pubblico ministero viene infatti richiesta non tanto la cultura della giurisdizione, ma la cultura dell'investigazione, tanto spesso trascurata. Al giudice, in ragione della sua posizione di terzietà imposta dalla Costituzione, si richiede quella imparzialità che tuteli le garanzie fondamentali dei cittadini. Anche a livello europeo - tanto invocato in altri momenti - è sufficiente un rapido esame per rendersi conto di come la disciplina di accesso e progressione in carriera sia differente rispetto a quella italiana. Ad esempio, in Germania si parte da un'unica formazione per tutte le professioni legali, che si articola in varie fasi e comprende esami di professionalità, al termine dei quali si sceglie una della professioni legali. A questo punto, giudici e pubblici ministeri godono di uno *status* giuridico distinto, che continua ad essere tale per tutta la progressione in carriera. Lo stesso dicasi per la Spagna, dove la carriera in magistratura è separata da quella di pubblico ministero. Si parte tuttavia da un concorso unico per giudici e pubblici ministeri, al termine del quale i vincitori scelgono tra una carriera e l'altra. Un altro risultato importante di questa riforma è la temporaneità degli incarichi direttivi (e ricordiamo a questo proposito che si tratta di un'antica rivendicazione della magistratura), oltre alla nuova strutturazione degli uffici della procura. La nuova previsione in chiave verticistica serve a recuperarne l'efficienza, individuando nel procuratore capo il compito di coordinamento della gestione delle indagini, ma serve anche a recuperare chiarezza, individuando il centro di responsabilità in colui che diventa l'unico titolare dell'azione penale. Con le modifiche realizzate siamo sicuri che, alla fine, gli uffici di procura recupereranno l'efficienza e l'agilità gestionale che sono troppo spesso mancate al procuratore nell'organizzare i lavori degli uffici a lui sottoposti. Condivisibile è anche la chiarezza con cui viene strutturato il sistema degli illeciti disciplinari che, in tal modo, dovrebbe finalmente diventare tassativo, chiaro e indirizzato al recupero dei valori di professionalità, equilibrio, correttezza, imparzialità, indipendenza: insomma, di quella che dovrebbe rappresentare l'autonomia vera, e non meramente proclamata, per l'esercizio della funzione giudiziaria. Riteniamo quindi che questa riforma sia stata varata, al di sopra degli interessi di parte, per rispondere ai problemi reali e contrastare l'inefficienza del sistema giustizia. E siamo convinti che, per poter fare questo, sia necessario creare un modello di magistrato più attuale e rispondente ai nuovi valori della moderna società società civile, per renderlo compatibile con la richiesta di giustizia del Paese e più rispondente ai principi costituzionali di imparzialità ed efficienza. A fronte di queste considerazioni, di cosa stiamo discutendo oggi? Della richiesta, da parte della maggioranza e del Governo, non di fare qualcosa al posto della legge comunque esistente con le caratteristiche che ho fin qui elencato, ma semplicemente di rinviare questa legge più avanti nel tempo, in attesa che l'attuale Governo, l'attuale maggioranza individuino una proposta alternativa e portino avanti una nuova proposta di legge. Devo dire che questa è un'abitudine abbastanza consolidata in questa maggioranza, che nei due anni precedenti le elezioni aveva fatto intendere al Paese di essere pronta a ribaltare l'Italia, a metterla a posto in tutti i suoi settori, salvo poi scoprire, dopo le elezioni, che in qualunque argomento si arrivi a discutere la posizione del Governo è semplicemente quella di attendere, di aspettare, di rinviare perché deve pensare cosa fare.

vaneggia su alcune proposte come quella dell'anno per ricerca di lavoro, quella dei ricongiungimenti facili, quella del certificato di famiglia dimostrato con una carta scritta a mano in qualche Paese del Terzo mondo, mentre in tutto il resto d'Europa anche Ministri competenti e Governi di sinistra vanno in direzione esattamente opposta, come lo stesso Prodi, che in casa dà ragione a Ferrero e poi va a stringere la mano a Zapatero che ha dichiarato che rimanderà a casa 800.000 immigrati.

molti di questi già rientrati in carcere, molti di questi che hanno commesso subito dopo la liberazione reati anche molto gravi, alcuni addirittura omicidi o lesioni gravi alle persone. Questo è il vostro modo di vedere la giustizia: criticare quello che con grande fatica e con grande sforzo è stato fatto da altri, cioè da noi nella scorsa legislatura, arrivando ad una legge, ripeto dopo cinquant'anni, che comunque ha una sua organicità e proponendo in cambio il nulla, se non di rinviare, mentre, devo dire, con molta velocità, siete riusciti a liberare 22.000 delinquenti. Tutto ciò serve a non far parlare e riflettere i rappresentanti del popolo, quali dovremmo essere noi, sugli effettivi problemi della giustizia. Ieri abbiamo sentito l'intervento del senatore D'Ambrosio, che, come giustamente ha ricordato il collega Fruscio, ha raccontato in maniera quasi suadente la situazione della magistratura, quasi come se raccontasse una favola ai nipotini di una magistratura che evidentemente conosce solo lui. Probabilmente non è più abituato a frequentare gli ambienti normali, dove vivono i cittadini normali, che non viaggiano con l'auto blu, la scorta,

guardiamo un attimo ai numeri. Dovremmo infatti governare il Paese anche dal punto di vista dell'utilizzo ottimale delle risorse, cioè delle tasse che i cittadini pagano con grande fatica. Ricordiamo i numeri: in Italia oltretutto con un aiuto che è stato dato: ho visto la richiesta delle associazioni dei magistrati fatta anche nella scorsa legislatura - abbiamo superato i 9.000 magistrati. Deteniamo il *record* mondiale di magistrati *pro capite*. Ricordo che la sola Campania ha un numero di magistrati equivalente a quello dell'intera Inghilterra. A fronte di ciò abbiamo quasi dieci milioni di processi civili in attesa di essere terminati e la durata media di tali processi è ormai vicina ai dieci anni di tempo. Ma sue queste cose i magistrati, le loro associazioni e i loro rappresentanti sindacali non hanno nulla da dire?

nell'espletamento dei processi? Perché nessuno parla qui della presenza dei magistrati? Hanno forse paura che magari al primo avviso di garanzia possano essere trattati peggio di altri? Io lo dico senza nessun problema (ho avuto la fortuna di non essere mai stato implicato in alcun processo anche per incarichi istituzionali che ho svolto nel passato, mi è accaduto spesso di assistere e di dover portare testimonianze). Perché nessuno parla, per esempio, di impegno fisico e di orario di lavoro dei magistrati? Perché non si fanno le statistiche rispetto agli altri Paesi europei ed occidentali su quanti giorni all'anno e quante ore al giorno

le procure o i tribunali non hanno i soldi per fare le fotocopie. Con tutti gli stipendi inutili che abbiamo nel sistema giustizia, ne faremmo non a milioni ma a miliardi di fotocopie! Ricordo, tra le altre cose, che i giudici

al cittadino non dovrebbe essere nascosto. Ci sono peraltro esempi che arrivano dal passato veramente eclatanti in questo senso, che solo con grande fatica sono stati Ricordiamo per esempio che, fino a una decina di anni fa (e proprio per intervento della Lega, all'inizio degli anni Novanta, tale scandalo fu eliminato, almeno questo, nel nostro Paese), i magistrati erano gli unici cittadini italiani che, se venivano eletti al Parlamento, continuavano a prendere lo stipendio da magistrato (potendo quindi disporre di un doppio stipendio, quello da magistrato e quello da parlamentare),

Una categoria di persone come loro, che hanno sindacati che si chiamano Magistratura Democratica, cioè che mettono nel nome del loro sindacato l'orientamento politico, come fa a dichiarare di essere oggettiva nel giudizio, soprattutto quando ad essere giudicate sono persone che hanno inevitabilmente un certo tipo di collocazione? Comunque, stavo dicendo che abbiamo avuto un fulgido esempio dal senatore D'Ambrosio, qualche settimana fa. Parlando dell'indulto,

Abbiamo visto la Forleo che scambia terroristi con guerriglieri (peraltro, se un guerrigliero fa il guerrigliero a casa mia, non vedo quale sia la differenza), che ha inveito contro i poliziotti perché avevano arrestato un soggetto che non aveva pagato il biglietto del tram, di essere incivili i poliziotti che con 1.200 euro al mese rischiano anche di prendersi quattro legnate da queste persone. Ma se nel Paese

quello definitivo dovrà essere, come nei Paesi seri e civili, l'elezione diretta del giudice. Una persona che vive fuori dal contesto e

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono passati 47 anni, dal gennaio 1948 al 25 luglio 2005, data in cui è stata approvata la legge delega per varare la riforma dell'ordinamento giudiziario, prevista dalla VII Disposizione transitoria della nostra Costituzione. È stato ridefinito l'esercizio dei poteri e delle funzioni all'interno dell'ordinamento giudiziario, con un forte scontro con l'Associazione nazionale dei magistrati e con l'opposizione del centro-sinistra.

che il clima di scontro in cui nacque e fu approvata la legge delega sulla riforma dell'ordinamento risentiva delle vicende processuali dell'allora Presidente del Consiglio e, quindi, muoveva da un «chiaro intento punitivo nei confronti della magistratura, la cui indipendenza - continua il collega D'Ambrosio - era considerata un pericolo». Riteniamo che un giudizio così pesante sia ingiusto nei confronti del Parlamento, ossia di quella maggioranza che votò la delega, tra cui il sottoscritto e l'UDC. Rassicuro il collega D'Ambrosio - e quanti la pensassero come lui - che non abbiamo mai avuto la preoccupazione delle vicende giudiziarie di Berlusconi; semmai, siamo stati preoccupati da una sconfitta del suo consenso popolare per via giudiziaria, ovvero da un uso strumentale del potere inquisitorio. Un altro autorevole collega dei Democratici di Sinistra, il senatore Calvi, intervenendo il 28 giugno 2006 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, pur affermando che si trattava di una legge pessima, ostile alla giurisdizione, di dubbia costituzionalità e lesiva dei principi di libertà ed uguaglianza, riconosceva che non vi era un conflitto tra Parlamento e magistratura, e che quindi la logica punitiva di cui parla D'Ambrosio è da riporre nella sua bellicosa fantasia. Non siamo così sprovveduti da ignorare che alcuni risentimenti e pregiudizi abbiano albeggiato nella volontà di alcuni parlamentari, ma non si può generalizzare al punto da invocare uno scontro, riassunto in quell'inno alla lotta delle toghe di Borrelli: «Resistere, resistere, resistere!». Il nostro Dio - come ha ben sostenuto Benedetto XVI - è quello della ragione e non abbiamo risposto alla dichiarazione di guerra di Borrelli. Sono amico personale di magistrati onesti, preparati e laboriosi. Noi dell'UDC non smetteremo mai di ricordare e riconoscere il tributo di sangue di magistrati eroici che hanno combattuto a fianco di quanti dei nostri esponenti, furono vittime del terrorismo tendente a scardinare lo Stato. Vi è una stragrande parte di magistrati che studia e lavora, che non teme i concorsi o qualunque forma di valutazione che non è vero che trascurerebbe di lavorare per ragioni di carriera. Vi sono giudici che non amano i colleghi procuratori in prima pagina, famosi nella fase dell'accusa, meno famosi, poi, in quella del giudizio, in cui troppe volte subiscono umilianti, quanto silenziose sconfitte, a nulla rilevando il dolore delle vittime. Il ministro Mastella ha ricordato ieri che l'ultima riforma dell'ordinamento risaliva al 1941: qualcuno avrà pur giudicato che era arrivata l'ora di riformare; probabilmente, qualche magistrato pensava di rimanere alla riforma Grandi del 1941; qualcun altro avrà pensato che la riscrittura dovesse essere realizzata a due mani: Associazione Nazionale Magistrati e Parlamento. Non sfugge però al presidente del Movimento per la difesa della Costituzione Scalfaro e a quanti l'hanno seguito per l'ultimo *referendum*, che la Costituzione va sempre difesa, anche quando la cultura della sovranità parlamentare incrocia maggioranze diverse dalla propria. Se questo è vero, dovete riconoscere che la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata votata in libertà, anche da chi, come me, riteneva fuori dal tempo la semplice laurea in giurisprudenza per l'accesso in magistratura che fosse arrivata l'ora di una sede specifica, come la Scuola Superiore della Magistratura, per una formazione permanente dei magistrati, così come avviene, in genere, per il lavoro privato e pubblico, e come ha sottolineato bene il presidente della Repubblica Napolitano alla sessione di insediamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura. Ci sarà pure chi è d'accordo con una separazione delle funzioni secondo una logica di valorizzazione delle proprie inclinazioni professionali. Non comprendiamo perché sulla separazione delle funzioni possano esprimersi autorevoli magistrati ed esponenti della sinistra e non abbiano diritto di farlo parlamentari del centro-destra. Non ho mai capito - e non lo hanno mai capito molti italiani - perché l'avanzamento economico e gerarchico nella magistratura fosse dettato dall'inesorabile invecchiamento di ciascuno e non dai meriti professionali, come in ogni luogo di lavoro del nostro Paese. Molti giovani magistrati - così come molti giovani farmacisti cari al ministro Bersani - non hanno mai capito perché la loro bravura e preparazione dovesse essere mortificata nell'accesso agli incarichi direttivi, semidirettivi e di legittimità dal privilegio di altri magistrati che opponevano la vecchiaia al merito. Non abbiamo capito - ma nemmeno molti capi delle procure italiane - come poter arginare il protagonismo mediatico e a volte anche l'arbitrio personale di alcuni sostituti procuratori che la precedente normativa rendeva liberi di accusare, dissacrare, sfigurare la dignità umana e professionale di chiunque incrociasse i loro pregiudizi o teoremi accusatori. Non abbiamo mai capito perché l'obbligatorietà dell'azione giudiziaria costituisse un *totem* sacrale della magistratura inquirente e la stessa volesse poi sottrarsi dalla stessa regola nei procedimenti disciplinari aperti dalla loro giustizia interna. Non ho mai capito perché un militante *no global* avesse dovuto credere all'imparzialità del giudice o al rinvio a giudizio di un sostituto procuratore dichiaratamente militante di AN o Forza Italia; ma il discorso vale con protagonisti invertiti. Ho votato la riforma Castelli per dare una risposta a questi interrogativi, miei e di milioni di italiani, molto più attratti da queste inquietudini che dalle supposte vendette di Berlusconi contro la magistratura. La domanda che c'è oggi in quest'Aula è se siamo riusciti in questo intento. Il ministro Mastella ha detto di sì. Nel suo discorso di ieri ha dichiarato che non vuole cancellare la riforma Castelli, perché non vuole realizzare né una controriforma, né una riforma diversa. Non so se parlava a titolo personale - come spesso gli capita - o a nome del Governo e della sua maggioranza; quindi a nome del senatore D'Ambrosio e del ministro Di Pietro. Sta di fatto che, rispetto ad un equilibrio politico possibile di riscrittura di alcune norme minori e di dettaglio, ha svolto un intervento da equilibrista, preoccupandosi di non scoprire quelle carte che una certa sinistra giudiziaria non gli avrebbe mai fatto giocare. Il problema è tutto su questo punto: ad un'opposizione pronta a discutere le innovazioni, peraltro minori, manca un interlocutore politico, nel Governo e nella maggioranza, credibile ed autorevole, con cui discutere e definire un decisivo percorso legislativo. Il ministro Mastella ha riconosciuto che le modifiche rispondono al criterio di essenzialità, ma non contraddicono i criteri ispiratori della riforma. In ordine all'accesso alla magistratura, è giusto quello che è stato scritto nella riforma, anzi rincara la dose nei requisiti, riconoscendo titoli perfino a chi è stato consigliere comunale, provinciale o regionale, oppure parlamentare. A tanta imprudenza nessuno di noi si era mai spinto; rinuncio a qualsiasi commento. Sulla dirompente questione della separazione delle funzioni, non solo il Ministro intende mantenere il principio della distinzione, reclamando però un consenso della maggioranza che non c'è, ma mantiene e rafforza le norme di procedura della riforma, chiedendo addirittura il parere dell'ordine degli avvocati: anche a questo riguardo nessuno di noi si era spinto a tale punto e mi astengo da ogni commento. L'unica pillola concessa ai radicali dell'Associazione nazionale magistrati, è l'abolizione della distinzione nell'accesso alla carriera di magistrato. Sulle progressioni di carriera, il Ministro propone l'abolizione di quello che era diventato un concorso per titoli per una valutazione quadriennale, comunque rinunciando al precedente automatismo. Bene la scuola superiore per la magistratura, bene l'ufficio del pubblico ministero, con qualche ritocco, bene la tipizzazione degli illeciti disciplinari, bene la neutralità politica, bene tutti gli altri istituti con qualche ritocco. Se così stanno le cose, perché non evitare la sospensione? O meglio: fatta salva l'essenza della riforma, si discuta subito delle modifiche tecniche da introdurre entro il 29 settembre 29 settembre e altre individuarle dopo, chiedendo, eventualmente, su queste disposizioni, la sospensione. Sentiamo su questo Parlamento, soprattutto su questo ramo del Senato, il peso e la responsabilità di una decisione. Concordo con chi ha sostenuto in quest'Aula, dalle fila del centro-sinistra, che la riforma dell'ordinamento deve avere al centro l'interesse del cittadino e non gli interessi di questa o quella parte politica; coloro che sostengono questa tesi devono però stare attenti a non sembrare i pretoriani di una corporazione. Un conto è chiedere la sospensione dei decreti-legislativi, perché ci sono dei meccanismi attuativi che ne rendono inapplicabili le disposizioni, un conto è sostenere la sospensione perché è scritto nel programma elettorale del centro-sinistra sotto dettatura della ANM. Se c'è l'onestà intellettuale di riconoscere l'interesse del cittadino, allora non si può avere la faziosità di individuarlo solo nella propria parte politica. Amici del centro-sinistra, abbiate il coraggio di abbandonare i vincoli del patto elettorale con un corrente politica militante della magistratura e accingetevi a riscrivere quelle norme che tecnicamente devono essere corrette o meglio calibrate, come ha ricordato il vice presidente del CSM Mancino. Noi dell'UDC, come ha ricordato il collega D'Onofrio, siamo pronti a farlo in piena autonomia e libertà di coscienza. La nostra opposizione non è contro il Paese, come spesso ci ricorda il collega Baccini, ma contro gli interessi di parte, qualunque essi siano.

«Occorre superare le tensioni tra politica e giustizia, inevitabilmente destinate a turbare lo svolgimento di una così alta funzione costituzionale»; «Il recupero di toni che non siano di pura contrapposizione agevola la ricerca di punti di convergenza ed evita che la dignità dei magistrati venga ingiustificatamente ferita da gratuite forme di delegittimazione»; «Il dialogo, inoltre, è premessa indispensabile per restituire funzionalità al sistema giustizia, essenziale servizio pubblico che, come tale, deve ispirarsi ai princìpi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione». Noi che siamo eredi del pensiero e della testimonianza di un uomo che la nostra storia repubblicana ricorda, come Bachelet, non possiamo non riconoscerci nelle parole del Capo dello Stato che ho citato.